che smentisce in modo clamoroso i dati diffusi dal Governo e dal ministro Fioroni in relazione ad alcuni aspetti importanti della finanziaria. Visto il ministro Fioroni aveva preannunciato il più grande piano di assunzioni nella storia della scuola italiana, mentre la realtà dei fatti sembrerebbe smentire clamorosamente tali affermazioni, chiedo che il Ministro venga invitato a riferire in Aula, perché francamente si tratterebbe di una bugia, di una menzogna

ha continuato con questa farsa dell'ipocrisia, dichiarando che in realtà i posti scoperti nei prossimi tre anni sarebbero di 150.000 unità, contando anche 42.000 posizioni che invece nella relazione tecnica del Governo vengono considerate già facenti parte di un complesso di posti vacanti pari a 116.000 unità.

per le assunzioni di personale precario. Siccome si tratta di una questione molto delicata, siccome dai dati in nostro possesso risulta che i posti disponibili per le assunzioni sono circa la metà o poco più di quanto preventivato dal Governo e siccome il Ministro continua invece ad insistere nel fornirci dati non corretti, chiedo che possa venire in Aula a rispondere con dati questa volta precisi.

L'incidente è avvenuto stamani alle ore 9,37 presso la stazione di piazza Vittorio della linea A della metropolitana. Un convoglio della metropolitana che era in arrivo alla stazione di piazza Vittorio ha tamponato il convoglio che sostava in quella stazione e che aveva già le porte aperte per la discesa e la salita dei passeggeri. Ad ora la situazione è di una vittima accertata, di una persona in condizioni molto gravi, sotto intervento chirurgico per sfondamento del torace, e un quadro di feriti, di cui 110 lievi,

Idue treni interessati dall'incidente fanno parte di una fornitura molto recente, entrata in esercizio dal 2005 in poi. Possiamo dire si tratti di convogli moderni

parlo di quelli ministeriali - non sono ancora arrivate ad alcuna conclusione circa le possibili cause. Posso fornire in questa seconda parte alcuni dati tecnici, che probabilmente non dicono molto, ma che credo siano comunque necessari per far capire in quale tipo di situazione l'impianto si trovasse. L'impianto di segnalamento della linea A ha la funzione di assicurare sia il distanziamento che la protezione dei treni in circolazione mediante un sistema chiamato ATP. Tale sistema è costituito da un impianto di blocco automatico per la trasmissione di informazioni di sicurezza ai treni e da apparati a bordo dei convogli per la ripetizione dei segnali, il controllo delle velocità e l'eventuale intervento della frenatura di soccorso del treno in caso di mancato intervento del macchinista. Provo a chiarire quanto detto, utilizzando termini più semplici. Ove il convoglio si trovi a percorrere una tratta per la quale è prevista una soglia di velocità, se la stessa in quel momento è superiore, c'è un avvisamento di natura acustica in cabina che dura sei secondi e che richiama l'attenzione del macchinista al fatto che deve frenare per portare la velocità sotto soglia. Se questo non avviene non avviene nei sei secondi, scatta un meccanismo automatico che frena il treno. Questo significa che dobbiamo pensare, ma vi prego di darmi conto del fatto che siamo alle prime considerazioni, che comunque la velocità del treno nel momento in cui è avvenuto il tamponamento dovesse essere abbastanza bassa, presumibilmente nell'ordine di 25-30 chilometri

fosse presente l'unica persona rimasta vittima, una giovane donna. Questo impianto di blocco - torno a dati di natura tecnica - consente la ripetizione continua dei segnali ed il controllo di velocità. Le informazioni trasmesse vengono captate da apposite bobine collocate in testa alle elettromotrici e sono trasformate in indicazioni luminose per il macchinista. Il dispositivo di bordo per il controllo della velocità confronta la velocità del veicolo con quella limite corrispondente al codice captato e il superamento della velocità limite provoca, in caso di mancato intervento del macchinista, come ho accennato prima, la frenatura del treno, che permane finché la velocità non torna al di sotto del limite. Il sistema di segnalamento di tipo continuo è integrato con uno discontinuo cui sono affidate funzioni di protezione in alcuni punti singolari. In prossimità di ogni segnale imperativo risulta sempre presente una duplice informazione di identificazione, che diventa operativa solo nel caso di mancato contemporaneo arrivo della trasmissione permissiva, cioè di via libera, per qualche situazione. Il convoglio di cui parliamo, oltre ad essere attrezzato con dispositivi che dialogano con sistemi di terra, è dotato di un dispositivo di arresto automatico che verifica la presenza attiva del macchinista, al fine di evitare situazioni di pericolo derivanti dalla perdita di controllo. Insomma, se per qualche ragione il macchinista avesse un malore

fatti collegati agli impianti di linea oppure a condizioni che in questo momento non possiamo sapere. Nulla, però, possiamo escludere perché - ripeto - si tratta di uno degli impianti tecnologicamente più avanzati, addirittura Per quanto riguarda l'attività del Ministero, sottolineo che ho già provveduto a nominare una commissione di inchiesta, presieduta dal direttore generale della sicurezza del trasporto del Ministero dei trasporti e composta da tecnici del settore e da un docente universitario esperto nel ramo.

Signor Presidente, a me spiace dover prendere la parola per problemi che riguardano Roma in una circostanza così drammatica;

non sa che si è intervenuti per quanto è stato possibile; anzi consiglierei di verificare se quella linea, allo stato, è in sicurezza

Veltroni e Rutelli, cioè Romolo e Remo, esserne i due figliocci, i due gemelli. Ho l'impressione che la storia sarà ricalcata anche per quello che conosciamo di Romolo e Remo.

I treni sono nuovi ma le tratte sono le stesse e siccome sono le stesse non possono essere allargate. Deve sapere, signor Ministro, che Dio ha voluto che l'incidente sia avvenuto in una stazione, perché se fosse accaduto - lo chieda al comandante dei Vigili del fuoco di Roma,

Chi conosce tali vicende sa dell'urgenza e della drammaticità di questi problemi, eppure abbiamo un'amministrazione che spende più per il Colosseo o per il Circo Massimo

di farci una relazione compiuta sulla linea A; non, però, su quello che si farà per Roma ma su quello che si è fatto per mettere in sicurezza la linea A della nostra capitale. In questo momento se mi dovessero ascoltare il prefetto di Roma, o chi lo ha preceduto, e il comandante dei Vigili del Fuoco, o chi lo ha preceduto, saprebbero bene di che sto parlando.

Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere venuto a informarci così tempestivamente, anche se le informazioni sono ancora molto poche. L'incidente è gravissimo e allo stato inspiegabile, quindi mi astengo da ogni ipotesi e da ogni giudizio che sarebbe assolutamente inadatto, visto che le conseguenze sono pesanti e il numero dei feriti elevato.

signor Ministro per la sensibilità e la tempestività con cui ha ritenuto di accogliere l'invito del presidente Marini.

sul quale fare e sviluppare i nostri ragionamenti. Penso che in questo momento il compito di chiedere il massimo rigore possibile per accertare se vi siano state responsabilità

funzionamento della commissione di inchiesta che lei già ci ha tempestivamente comunicato di aver insediato, soprattutto in ordine alle cose cui faceva riferimento il senatore Cutrufo. Per quanto riguarda la messa in sicurezza, troppe volte siamo costretti ad ascoltare dagli operatori del settore che probabilmente, sotto questo aspetto, qualcosa non funziona nei nostri trasporti. Credo che sia necessario il massimo rigore, soprattutto sotto questo profilo; è bene che lei riceva le sollecitazioni su questi aspetti da chi in questo Parlamento le ha dato la fiducia e in questo momento le chiede di applicare, al di là delle appartenenze, il massimo rigore nella verifica dell'evento e, soprattutto, nella prevenzione. Noi vorremmo, signor Ministro, colleghi dell'Aula, non doverci trovare altre volte a ragionare sulla base di un evento increscioso, brutto e tragico come quello di stamattina. Vorremmo invece ragionare di altre cose, di come fare per evitare che tali eventi

quindi buon lavoro alla commissione di inchiesta ed esprimo solidarietà a coloro che ancora sono in situazioni sanitarie precarie. Ci auguriamo che la stessa commissione non ci debba far riconsiderare acquisti fatti recentemente; dalla sua relazione, signor Ministro, ci è infatti sembrato di capire che dovremmo essere all'avanguardia della tecnologia in termini di sicurezza. Purtroppo, nel caso di specie, così non è stato. La preghiamo di tenerci costantemente informati proprio per realizzare un momento di prevenzione che sia cosa diversa dal celebrare un evento tragico. Signor Presidente, anche da parte del Gruppo della Lega Nord desidero esprimere alla famiglia della vittima - speriamo sia l'unica

sui sistemi di sicurezza di questi impianti, che, se mi permette, evidentemente lasciano molto a desiderare. Ci ha anche detto che li esportiamo all'estero: speriamo non ci facciano fare brutte figure.

a parte il fatto che senz'altro le scatole nere forniranno informazioni assolutamente dettagliate sull'accaduto, siamo nel 2006, signor Ministro, e penso che certi sistemi di sicurezza possano essere veramente attivati per la sicurezza di tutti, soprattutto soprattutto di quei pendolari che vengono nella capitale quotidianamente per lavorare. Colgo l'occasione per sollecitare a lei,

Signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo dell'UDC esprime un sentimento di cordoglio autentico e anche di dolore verso le famiglie colpite da questo gravissimo incidente.

capitale, riscopre due autentiche problematiche; una l'abbiamo ascoltata dal Ministro competente, ed è la problematica di carattere tecnico, di come possa essere avvenuto, nell'era della tecnologia, un incidente di così elevata gravità. Abbiamo sentito dal Ministro le considerazioni sulla nuova tecnologia e abbiamo appreso che questi treni sono stati addirittura acquistati dal Comune di Roma recentemente; altri colleghi hanno posto, signor Ministro, il problema delle infrastrutture e se risponde a verità - e questo è l'interrogativo che lasciamo alla sua autorevole valutazione di Ministro competente che la distrazione di risorse nella città di Roma abbia impedito in termini di priorità le manutenzioni necessarie e la messa in sicurezza degli impianti, non solo delle metropolitane, ma del comparto dei trasporti e della viabilità in generale. Signor Ministro, questi sono problemi sicuramente tecnici; aspettiamo la commissione d'inchiesta ministeriale e vogliamo chiedere alla Presidenza del Senato di valutare l'opportunità di aprire un'inchiesta parlamentare conoscitiva sull'evento e la questione romana. Non voglio toccare, per ovvie ragioni, argomenti più specifici sulle responsabilità politiche lo faremo in un'altra sede, non in questa seduta di cordoglio e di apprensione - ma sicuramente non possiamo tacere, in un'Aula e in un consesso così importante e autorevole, anche le responsabilità politiche. Signor Ministro, ella sa, essendo un tecnico e un universitario di rango, che quando esiste un problema tecnico a monte c'è sempre una responsabilità politica. Vorremmo chiedere a lei, perché lo chiedono le famiglie, lo chiedono i lavoratori di Roma, delle metropolitane, che non avvenga anche in quest'occasione l'insabbiatura delle responsabilità. vorrei infatti che fossero i soliti a pagare (perché di questo stiamo parlando): noi vogliamo sapere i nomi e i cognomi dei responsabili sia dal punto di vista tecnico sia, soprattutto, dal punto di vista politico. Non vorrei che fosse il solito ferroviere - magari ricorrendo alla classica citazione dell'errore umano - a farsi carico della completa responsabilità del fatto. Sono convinto che esistono agli atti dell'amministrazione comunale numerose segnalazioni, e lei può accertare, signor Ministro, se a Roma è stato omesso di dare seguito a segnalazioni di perdite di acqua durante il percorso della linea A; se inoltre - e ho concluso, signor Presidente - vi sono responsabilità politiche sulla mancata manutenzione degli impianti

che il sindaco di Roma, al quale va tutto il nostro riconoscimento per quello che sta facendo, crei l'ennesima commissione per scaricare le responsabilità - che sono sue dal punto di vista politico sull'universo mondo della responsabilità amministrativa. Il sindaco è il capo dell'amministrazione, il sindaco ha comprato questi treni, il sindaco doveva fare le manutenzioni degli impianti e il sindaco dovrà rispondere a Roma e all'Italia di quest'ennesimo incidente nella nostra città.

Ovviamente da parte nostra, da parte del Gruppo di Rifondazione Comunista, si esprime tutto il cordoglio per la giovane lavoratrice morta e la solidarietà e la vicinanza ai feriti e alle famiglie di tutti quanti sono stati colpiti. Credo che sia anche giusto e doveroso esprimere un plauso alle forze che hanno, come tutti riconoscono, operato nel pronto intervento, dai vigili urbani ai vigili del fuoco, alla polizia, ai carabinieri, al personale sanitario, e una solidarietà alla città di Roma, che è indubbiamente colpita da un evento così grave. Penso che, al di là delle strumentalizzazioni politiche, che forse davvero non hanno senso in questo momento, sia da accertare con molta attenzione la causa di questo incidente, perché è davvero grave che apparecchiature come quelle da lei descritte, abbiano potuto determinare un incidente come quello che è avvenuto. I ferrovieri conoscono bene

sicché, anche nel caso di malessere, qualora il peso sul pedale venisse meno scatterebbe il meccanismo d'emergenza e quindi anche il blocco. I ferrovieri, però, hanno sempre denunciato questo meccanismo perché non è dato agli ingegneri progettisti conoscere le modalità del malessere eventuale del macchinista che si trovasse ad agire su quel meccanismo e da questo punto di vista occorre davvero essere molto attenti e molto rigorosi. Credo sarebbe bene che un'eventuale Commissione d'inchiesta di tipo parlamentare fosse rivolta, forse anche a partire dal drammatico incidente di oggi, a svolgere un'indagine sul sistema dei trasporti pubblici locali, sul loro stato di ammodernamento, sul loro stato di funzionamento, sul loro grado di finanziamento in questi anni, sul loro grado di sviluppo, sulle determinazioni che Aspettiamo davvero l'esito delle inchieste: c'è una commissione ministeriale che ha annunciato il Ministro; c'è l'indagine della magistratura, che ovviamente si avvarrà delle competenze tecniche; ci saranno certamente le indagini e le valutazioni da parte dell'azienda e da parte dell'amministrazione. Vorrei che, oltre agli aspetti tecnici,

perché molto spesso questo elemento incide. Soprattutto, vorrei che l'indagine ministeriale non si soffermasse esclusivamente sull'incidente, ma si estendesse allo stato di esercizio dell'intera rete, anche perché i dati i dati che lasciano intendere che nella rete ci fosse un ripetersi di segnali e di elementi di disfunzione

siamo in una sede parlamentare e credo che non vada nascosto nulla. A me fa piacere che i colleghi del centro-sinistra ringrazino il ministro Bianchi per la sua tempestività. Io non ritengo di doverlo ringraziare, perché ho l'impressione che quella che è una tragedia l'abbia considerata un atto formale nel suo racconto al Parlamento. Vede, Ministro, noi abbiamo la morte nel cuore perché una giovane pendolare, che veniva da una terra che ha dato molti morti al lavoro, la Ciociaria, oggi ha concluso la sua esistenza a causa di qualcuno che fa male i conti ogni volta che si tratta di metter mano al servizio pubblico chiamato trasporto locale.

Purtroppo dalla sua voce non abbiamo ascoltato nulla di tutto ciò. Lei, ed è apprezzabile, ha annunciato l'iniziativa di costituire una commissione ministeriale; ciò che non è apprezzabile è che non ci dica nulla sui tempi che ha dato a questa commissione e su quali competenze intende intervenire il Ministero in tema di sicurezza della metropolitana. Vede, Ministro, le responsabilità e i responsabili, come diceva il collega Baccini, ci sono, eccome! Sui *mass media* ci sono nomi e cognomi di quanti hanno colpevolmente trascurato il dramma della metropolitana di Roma. Le voglio ricordare che questa storia comincia da lontano. È agli atti del Parlamento un'interrogazione del senatore Menardi, di Alleanza Nazionale, persino sulla gara che ha visto consegnare alla società, della quale lei ha avuto il buon gusto di non fare il nome, la CAF spagnola,

questa mattina, dopo la tragedia che poteva provocare una vera e propria strage (parliamo di 110 feriti e per questo abbiamo chiesto la presenza del Governo in Aula), ha confermato che si tratta di uno dei nuovi treni CAF spagnoli,

Vittorio Emanuale, Repubblica, Barberini e Spagna», dal nome delle stazioni della metropolitana di Roma. Chi è che deve ammodernare? Chi è che non risponde all'appello del presidente di questa società che gestisce la metropolitana di Roma? Non è la prima volta che emerge questo scandalo. Nell'aprile 2005, proprio quando sono state collaudate le strutture che oggi sono state tristemente protagoniste di questo incidente (parlo dei vagoni dell'azienda spagnola CAF), un treno metro vuoto ha urtato con i respingenti nel deposito in prova nuovi convogli.

li mettiamo in conto e ci consentono ulteriormente di testare i nuovi mezzi. I nuovi treni devono circolare per due anni senza viaggiatori lungo circuiti predisposti fuori dalle linee e affrontare prove durissime. Questo serve a mettere i treni in condizioni di massima sicurezza». ancora: il sindaco Veltroni chiede due anni dopo di garantire sicurezza ai passeggeri. Questo accade quando i buoi sono scappati, quando le tragedie sono avvenute, nonostante fossero state annunciate. Signor Ministro, signor Presidente, dicendo che siamo stanchi di dover piangere dei morti perché nessuno interviene quando l'allarme viene lanciato. In questa città trascorriamo una volta l'anno una notte bianca, ma ci sono ancora 365 giorni neri. Meno feste e più servizi.

dal senatore Storace - non si può non evidenziare il grande lavoro messo in atto nelle operazioni di soccorso (che ha sicuramente limitato gli effetti dell'incidente) da parte della Polizia, dei vigili urbani, dei Vigili del fuoco e dei cittadini romani che hanno immediatamente solidarizzato con chi era stato incidentato. Questo, però,

Met.Ro: nei vecchi treni la frenata dava più sicurezza a chi guidava. Chi conduce invece il treno CAF deve mantenere un livello di attenzione ben superiore al normale. A ciò aggiungono una denuncia, veramente molto seria e grave:

Ancora: nell'ultima settimana, cari colleghi, dal 9 al 16 ottobre, ci sono stati circa 40 guasti sulla linea A, che hanno riguardato anche i nuovi convogli CAF.

Noi chiediamo al Governo di continuare con decisione su questa stessa impostazione. Come non ricordare che noi abbiamo approvato un nuovo organismo per la sicurezza ferroviaria? Chiediamo al Ministro di attuarlo. La scorsa finanziaria ha visto nascere l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Sono state annunciate dall'ANSA tre diverse commissioni di inchiesta: la sua, signor Ministro, quella del Presidente Marrazzo e, infine, quella del sindaco Veltroni, oltre che, naturalmente, quella della magistratura. Non vorremmo che le commissioni d'inchiesta fossero funzionali a chi le fa. Al contrario, l'esistenza di un'Agenzia per la sicurezza ferroviaria consentirebbe a un ente terzo

anche noi, come Ulivo, siamo vicini ai parenti della vittima

È come se noi - caro senatore Storace - nei cinque anni passati, dal 2001 al 2005, strumentalizzato e chiamato in causa il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro dei trasporti, allora senatore Lunardi, quando nel sistema ferroviario italiano abbiamo avuto ben 69 incidenti,

che chiamava in causa sicuramente un problema che riguarda la sicurezza delle nostre linee e del nostro armamento ferroviario! STORACE *(AN)*. Abbiamo compiuto una scelta completamente diversa, che è quella di tener conto dell'incidente grave che vi è stato. Per lo meno questa sera, pensavo che i colleghi dell'opposizione facessero altrettanto, di fronte ad un incidente come quello romano, invece no:

e che, solo negli ultimi tre anni, si sono spesi nelle stazioni e nel sistema della sicurezza ben 200 milioni di euro e che altri 300 milioni di euro sono stati spesi per

Certo, potevamo fare di più. Credo che l'amministrazione comunale potesse fare sicuramente molto di più rispetto a quello che ha fatto, ma a una condizione:

nel sistema ferroviario e metropolitano. Purtroppo qualcuno dimentica che, soprattutto nelle ultime finanziarie, c'è stato un taglio netto nell'intervento sulle ferrovie, sulle metropolitane e, in particolare, sul trasporto pubblico locale.

e chiama in causa il centro-destra che ha fatto altrettanto appunto nei confronti degli enti locali e del Comune di Roma.

Signor Presidente,

cui dobbiamo fornire risposte; altrimenti rischiamo di trovarci in un prossimo futuro a piangere nuovi morti. Già troppo spesso questo è accaduto. I dubbi riguardano diversi aspetti: l'aspetto economico, a proposito dei costi, l'aspetto delle regole, assolutamente incerte, ed il quadro politico, mutato in maniera drammatica, repentina e probabilmente neanche prevista, da agosto ad oggi. Sui costi - se mi permette - vado velocemente. Ci apprestiamo ad esaminare una legge finanziaria che prevede più tasse. Sarebbe sicuramente meglio spendere i soldi, che sono pochi, all'interno del Paese, piuttosto che in missioni all'estero che oggi non hanno più una certezza, come qualche mese fa. Per quanto riguarda le regole, ci stupisce questa mancanza di chiarezza sulle cosiddette regole di ingaggio, termine che ormai è diventato di uso comune. Si è detto tutto e il contrario di tutto e sarebbe bene sapere in modo definitivo che cosa ne pensino davvero all'interno di questo Parlamento. Un conto è dire «andiamo a compiere un'azione di pace», altro è dire «interveniamo per fare da cuscinetto tra Israele ed il Libano». Credo che la maggior parte di voi - almeno lo spero - abbia letto il libro molto bello di Oriana Fallaci «Insciallah», che racconta la realtà della «polveriera Libano». Se vogliamo, erano tempi più semplici di quelli attuali. Un cittadino delle mie parti che ha partecipato a quella missione mi ha raccontato che all'epoca è andato tutto bene anche perché la missione dell'esercito è stata molto più semplice: sono arrivati in Libano e si sono chiusi nei *bunker*. frattempo, la nave che doveva riportarli ha subìto un ritardo). Adesso non è così. Adesso stiamo andando in Libano con l'avallo della sinistra radicale (la stessa che fino a qualche mese fa si dichiarava pacifista e contraria ad ogni intervento armato; sarebbe bello capire la logica di certi atteggiamenti), ma non si capisce bene perché, per come e per fare un favore a chi. L'impressione è che la missione sia sempre più sbilanciata pro Libano, contro il cattivo Israele che ha un brutto vizio, signor Presidente: di difendersi quando lo bombardano. Notiamo un'ipocrisia pacifista, se mi permette, a questo riguardo, che si è manifestata anche stamattina per bocca del collega senatore Grassi di Rifondazione Comunista, che quando non ha argomenti insulta la Lega Nord e suoi esponenti, dandoci degli xenofobi, dei razzisti e quant'altro: questo dimostra una pochezza intellettuale che si commenta da sola. Al di là dell'ipocrisia pacifista, che però non stupisce più di tanto, perché sappiamo che questo Governo oramai tiene tutti insieme con lo *scotch*, aspettando forse un nuovo Governo, al di là di questi aspetti contingenti, non si scherza, signor Presidente, sulla pelle dei nostri ragazzi. Non possiamo trovarci ogni volta a dover piangere i morti senza sapere perché e percome mandiamo i nostri ragazzi all'estero. A questo punto, non possiamo fare altro che porci dei dubbi, è nostro dovere porci dei dubbi: ha senso, in uno scenario che è mutato in maniera così repentina e drammatica, la missione così come è stata impostata inizialmente? Ha senso che non si sappia esattamente quali sono i poteri di reazione dei nostri militari? Ha senso buttare una marea di soldi, e non si sa quanti, quando di soldi ne abbiamo pochi per risolvere i nostri problemi interni? Non è forse meglio pensarci bene, signor Presidente, pensarci dieci, cento, mille volte (parafrasando un'affermazione dei pacifisti *no global*, amici di una buona parte di questo Parlamento)? Pensiamoci dieci, cento, mille volte prima di mandare allo sbaraglio i nostri ragazzi, per evitare di doverci trovare ancora a dover piangere dei morti non si sa bene perché e per colpa di chi.

colleghi, la senatrice Alberti Casellati stamani si domandava dove sono i pacifisti. Vorrei sommessamente dire alla senatrice che se si volta da questa parte troverà dei pacifisti. Spero, va da sé, che trovi pacifisti anche in altre componenti politiche, perché perché mi pare un' esigenza che abbiamo tutti, che ha il Parlamento italiano, che ha il popolo italiano, quella di lavorare perché siano in qualche modo messi sotto osservazione perlomeno i punti più drammatici delle crisi nel mondo. Ho anche sentito il senatore Tonini, di cui ho apprezzato l'intervento, parlare e stabilire una distinzione nel pacifismo: ci sarebbe infatti un pacifismo buono, quello non isolazionista. Vorrei dire al senatore Tonini che il pacifismo per essere tale non può, direi per statuto, essere isolazionista. Questo vale oggi di fronte alla guerra globale, ai processi che sono all'ordine del giorno nel mondo e soprattutto nei punti di maggiore crisi, ma era vero anche in altri tempi. Il senatore Tonini, buon per lui, è molto più giovane di me, che quando il movimento pacifista italiano appunto protestava e marciava contro la guerra in Vietnam, questo veniva fatto anche a Washington, a Berkeley, a Parigi, a Roma e a Firenze. Ricordo appunto - io che sono più anziano del senatore Tonini - una grande manifestazione internazionale degli studenti universitari a Firenze. Mi pare che la frase che sosteneva questa manifestazione fosse quella di Tacito; se ricordo bene diceva su per giù: «Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato pace». Allora, mi pare che questo sia un impegno che dobbiamo mantenere nel nostro DNA di forze progressiste e di sinistra. La seconda questione che vorrei richiamare alla vostra attenzione è la caratteristica di questa missione. Capisco bene che ci sia uno sforzo per altro assolutamente destituito di fondamento per stabilire una connessione

dei rapporti geopolitici all'interno di un'area così delicata come quella del Medio Oriente e anche - questa è l'ambizione di maggiore portata - la possibilità di rimuovere le cause strutturali del conflitto. Altrettanto francamente

cari colleghi e colleghe, che la materia sia così rilevante che francamente non meriterebbe una riduzione a mero contenzioso politico a fini assolutamente interni,

con il pensiero che si tratta di una missione - come ha ricordato mi pare onestamente il ministro Parisi - lunga, impegnativa, costosa - anche se è quello che in questa fase m'interessa e ci dovrebbe interessare di meno - e rischiosa.

del Parlamento. Quindi, non pensiamo che sia il ballo dell'hotel Excelsior, ma sosteniamo - e chiudo, signor Presidente - che c'è stato un salto, che c'è un elemento di discontinuità che non vale una volta per tutte. Sappiamo che noi, come forza della sinistra più radicale, come veniamo definiti, dobbiamo mantenere la nostra vigilanza rispetto a questa discontinuità

Assimilare tutto alle forze terroristiche, alla rete di Al Qaeda, non ci aiuta ad individuare invece all'interno di quelle stesse forze quali siano gli elementi che possiamo mettere in corsa, che possiamo accelerare, su cui possiamo lavorare perché finalmente si risolva in quella zona il problema dei problemi: l'esistenza di due Stati, due popoli, uno palestinese e l'altro israeliano.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi riconosco totalmente nell'intervento del presidente De Gregorio, questa mattina, ha sostituito il senatore Ramponi, relatore, al quale anch'io formulo i migliori auguri per una pronta guarigione. Le polemiche e i distinguo che accompagnarono l'inizio dell'*iter* di conversione di questo decreto-legge alla Camera erano indubbiamente anche legati al fatto che, da parte di alcuni ambienti dell'attuale maggioranza, si voleva strumentalmente distinguere la missione in Libano dalle altre, segnatamente da quelle in Afghanistan e in Iraq, presentando la prima come vera missione di pace e le altre invece come missioni di guerra deliberate quasi in spregio dell'articolo 11 della Costituzione. Dal sacrificio dei nostri tredici aviatori a Kindu, in occasione della nostra prima missione dopo la fine del secondo conflitto mondiale, alle altre in Somalia, in Mozambico, nella ex Jugoslavia, con Kosovo e Bosnia-Erzegovina, in Afghanistan e in Iraq, Iraq, tutte le nostre missioni sono sempre state di pace, sia che fossero di *peacekeeping* che di *peace-enforcing*. In quelle lontane regioni abbiamo costruito o ricostruito ospedali, scuole, ponti, strade, ferrovie, infrastrutture con il nostro Genio militare. In Iraq abbiamo reso autonome le forze di sicurezza. Sempre e comunque missioni di pace con i nostri soldati per garantire alle varie popolazioni pace nella sicurezza, che è proprio ciò che ci chiedevano. Missioni di pace anche quelle disposte dal precedente Governo di centro-sinistra, alle quali non abbiamo fatto mancare il sostegno. Missioni di pace con i nostri militari armati. Mai, dico mai, abbiamo mandato solo i nostri cappellani, solo le nostre suore, solo le nostre crocerossine. Neanche in questa missione lo facciamo. Alla Camera il Governo, da noi sollecitato, di pace - ripeto, tutte le nostre missioni di pace - sono state disposte nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione. Missione di pace dunque anche questa in Libano. Missioni di pace tutte le altre, comprese quelle in Afghanistan e in Iraq. In questa occasione notiamo anche noi che non sventolano più le bandiere arcobaleno. Anzi, sono totalmente, o quasi, scomparse. Dove sono finiti, onorevoli senatori, gli sbandieratori? Se essi sventolavano davvero per la pace, perché non sventolano più? Di pace nel Medio Oriente e nel mondo c'era bisogno ieri, ieri, come c'è bisogno oggi, allo stesso modo. La verità è che gli sventolatori di professione sventolavano le bandiere arcobaleno non per la pace, ma contro il Governo Berlusconi. Questa è la verità. Il Governo Berlusconi era accusato di essere guerrafondaio, di operare in violazione della nostra Costituzione. Prendiamo comunque atto che gli sbandieratori non sventolano più. Però se fossimo stati noi oggi al Governo, onorevole Presidente, e se avessimo mandato noi in Libano migliaia di nostri militari, gli sbandieratori di professione cosa avrebbero fatto? Cosa avrebbe fatto la sinistra cosiddetta radicale, e non solo lei? Cosa sarebbe successo nelle piazze e in questa stessa Aula? Cosa avrebbe fatto il sindacato, sempre pronto a mobilitarsi per ragioni politiche e quasi mai per tutelare veramente i lavoratori di oggi e, soprattutto, quelli di domani? Quanti emendamenti e quanti ordini del giorno sarebbero stati presentati? Oggi nessuno o quasi. l'importante è garantire il pieno appoggio del Parlamento ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze con le stellette in una missione difficile e gravida di rischi, che non può e non deve essere affrontata con troppa enfasi e poca serietà. ragazze e ragazzi che hanno sempre portato con onore e con amore la nostra bandiera, il Tricolore d'Italia; ragazze e ragazzi che in Libano dovranno essere forza di interposizione fra i militari di Israele e gli Hezbollah, ben sapendo che questi ultimi vogliono da sempre l'eliminazione fisica dello Stato di Israele. In Libano dobbiamo favorire il disarmo di Hezbollah,

Il nostro sì, quindi, è condizionato agli sviluppi che avrà la missione perché non vogliamo, né direttamente né indirettamente, né oggi né domani, essere complici di terroristi assassini né in qualsiasi modo favorirli.

Signor Presidente, signori senatori, signori del Governo, con un voto di larga maggioranza che valica lo spartiacque fra il Governo e l'opposizione, il Senato si appresta a convertire in legge il decreto sulla missione militare in Libano, intrapresa in conformità alla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. La spedizione in corso ufficialmente (il senatore Sterpa direbbe «formalmente») è una prosecuzione rafforzata della missione UNIFIL che dura dal 1978, costata ai contingenti delle Nazioni Unite il sacrificio di molti soldati (come ha ricordato stamani, tra gli altri, il senatore Guzzanti). Peraltro, non è valsa a conseguire i risultati voluti, tanto che ancora a luglio l'osservatorio strategico del centro di studi militari definiva l'UNIFIL «il contingente dimenticato». La nuova missione comporta responsabilità che la storia non potrà, invece, in alcun caso dimenticare. I rischi e le difficoltà dell'impresa sono tali da sconsigliare i toni del trionfalismo; le sue ragioni inducono, come di fatto è avvenuto nel dibattito parlamentare, a guardare al di là delle visioni di parte. A scansare i toni del trionfalismo è stato anzitutto, nei lavori delle Commissioni, il Ministro della difesa: Arturo Parisi ha parlato di una missione lunga, impegnativa, costosa, rischiosa ed insieme doverosa, giusta ed urgente.

Sarà una missione lunga se solo si consideri che la prima UNIFIL è durata quasi 30 anni come missione *ad interim*; sarà costosa per le Forze armate italiane, storicamente sottocapitalizzate da uno squilibrio negli investimenti cui soltanto adesso, con il disegno di legge finanziaria di prossima discussione, si comincia a porre parziale rimedio; sarà - lo ammonisce la dichiarazione di voto distribuita in anticipo stamani dal senatore Cossiga - inevitabilmente rischiosa, data la cronica instabilità dell'area in cui l'UNIFIL ha il mandato non solo di schierarsi per interposizione, ma di impedire che avvengano operazioni ostili di alcun tipo; sarà, infine, impegnativa perché in Libano non c'è una pace, ma per ora c'è soltanto una tregua ed il mantenimento della tregua dipende non soltanto dal debole Governo libanese, ma dalle pressioni della Siria e dell'Iran. Il mandato della risoluzione 1701 ha per obiettivo principale il ripristino della sovranità del Governo libanese di cui è parte anche il movimento degli Hezbollah, cui la stessa risoluzione delle Nazioni Unite attribuisce l'inizio delle ostilità; è del tutto imprevedibile cosa il Governo libanese potrà fare per disarmare le milizie irregolari e per garantire che almeno nella zona di confine siano presenti soltanto le armi autorizzate. Va dato atto al Governo israeliano di aver accettato un criterio realistico, quale è comunque preferibile negoziare con un Governo piuttosto che dover fare i conti con l'anarchia. Ma certamente la soluzione della conflittualità resta consegnata ad un futuro di lungo termine. A fronte delle difficoltà e dei rischi stanno le ragioni della responsabilità di primo piano che l'Italia è chiamata ad assumere in forza della sua collocazione geopolitica e del suo ruolo specifico nel Mediterraneo. Sono, anzi erano, ragioni urgenti, visto che l'impegno prodigato dal Governo italiano è valso già, quanto meno, a fermare il massacro e ad assicurare la tregua (su questo almeno anche il senatore Guzzanti è d'accordo). E sono soprattutto ragioni giuste, intanto perché la spedizione è stata sollecitata da entrambi gli Stati contendenti e poi perché la partecipazione di militari europei a fianco di Stati islamici e anche della Cina lascia intravedere un futuro in cui allo scontro fra civiltà si sostituisca la volontà internazionale di pacificazione, la volontà di agire per porre termine all'interminabile conflitto fra Israele, Palestina e Siria e di arrivare (chissà quando!) a risolvere quella conflittualità che dell'instabilità mediorientale è insieme la madre e anche la figlia. Essendo queste le ragioni dell'iniziativa italiana è apprezzabile che nel dibattito sulla conversione in legge del decreto si sia posto termine alle polemiche retrospettive per stabilire una larga convergenza a sostegno dell'organizzazione delle Nazioni Unite quale necessario protagonista di un multilateralismo efficace. Signori senatori, una politica internazionale di multilateralismo efficace richiama l'Unione Europea alla costruzione della politica comune della sicurezza e della difesa che il trattato costituzionale tuttora incompiuto esplicitamente vincola ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed agli obblighi derivanti dall'Alleanza atlantica. Se il processo costituente europeo non si fosse disgraziatamente inceppato, l'Unione avrebbe potuto essere presente in Libano in forme più dirette rispetto alla presenza dei contingenti nazionali dei suoi maggiori Stati membri. Ma va dato atto al Governo italiano, e segnatamente all'azione esercitata dal ministro degli affari esteri Massimo D'Alema, di non aver tralasciato ogni iniziativa utile per europeizzare la missione in Libano. La trama stessa della risoluzione 1701 sta nelle conclusioni della Conferenza internazionale riunita a Roma il 27 luglio, con la partecipazione, insieme alle Nazioni Unite ed a 14 Governi, di cui la metà europei, delle istituzioni dell'Unione (l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Presidenza di turno finlandese, la Commissione). L'attuazione risoluzione della 1701 è impegno comune dell'Unione fin dal 25 agosto E' essenziale che l'Europa, come è stato detto, decida una buona volta di andare oltre la funzione di ufficiale pagatore per assumere quella di attore strategico nell'area più decisiva per la propria sicurezza e per la costruzione della pace. Ciò sarebbe possibile nei fatti e non soltanto a parole se l'Unione disponesse della forza di intervento rapido programmata fin dal 1999 e di cui avrebbe dovuto dotarsi fin dal 2003. Abbiamo tutti in mente cosa ha detto in proposito, nel discorso di Trento per il premio De Gasperi, il presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La sua irriducibile fede europeista e quella del suo successore, Giorgio Napolitano, indicano la strada diritta che l'Italia deve seguire

e per senso di responsabilità nei confronti dei nostri soldati, noi voteremo sì a questo provvedimento. Riteniamo, però, che nella storia d'Italia sono scritti i motivi di diversificazione, anche profonda, che motivano il sì della maggioranza rispetto al sì di parte consistente dell'opposizione. Signor Presidente, la nostra politica estera si è sempre imperniata su tre capisaldi: Nazioni Unite, filoatlantismo ed Unione Europea. Ma vi sono stati modi diversi di interpretare questi tre capisaldi. Vi è stata una diversificazione sottile, che ha attraversato tutta quanta la storia dell'Italia, sin dalla nascita della Repubblica. Perché,

...una posizione filosovietica, dicevo, espressa in particolar modo dalle sinistre, e una posizione neutralista, che all'inizio e per un lungo periodo, fino agli inizi degli anni Cinquanta, ha avuto una sua plausibilità. Lo stesso modo di interpretare l'europeismo, all'interno della nostra storia, non è stato univoco; vi è stato chi ha ritenuto che l'europeismo fosse la declinazione obbligatoria dell'atlantismo e che significasse l'unione delle due sponde dell'Atlantico nei valori di una medesima civiltà e chi ha interpretato invece l'europeismo come il surrogato di quel neutralismo che non si poteva più sostenere nel momento nel quale la guerra fredda andava consolidandosi e il bipolarismo si trasformava nella struttura che sosteneva l'equilibrio planetario. Allora,

ma è altrettanto evidente che questa dialettica la ritroviamo oggi in questa Aula: nei due modi diversi di dire sì a questo

intervento proprio in quell'area geopolitica che oggi è interessata dalla missione di cui stiamo parlando. Fu un tentativo importante che trova posto tra le grandi pagine della nostra politica estera, ma fu un tentativo velleitario che finì male, che durò lo spazio di un giorno; bastò che la Francia riprendesse il suo ruolo nella zona dopo il 1958, e ancora di più dopo il 1962, e la parentesi

quando la nostra funzione si sarebbe potuta compiutamente svolgere attraverso un utilizzo e un'esposizione più modesta? Era necessario, dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista scenografico, rinverdire il mito della grande proletaria che abbiamo sentito echeggiare nell'intervento del Presidente del Consiglio, a bordo di una nave che non era ancora andata? Era necessario attribuire ad un'organizzazione terroristica la dignità di partito politico? Era necessario farsi prendere sotto braccio da un esponente di Hezbollah? Signor Presidente, ho l'impressione che tutto ciò era necessario; era necessario per riunire su una linea che avesse dignità di politica estera una maggioranza nella quale si muovono invece

dove l'ambizione di prendere la testa di una politica estera europea ha portato a delle esagerazioni in nome di una politica estera che in realtà non c'è: l'abbiamo sentito da ultimo anche nell'intervento del collega Zanone. La Francia ha reagito per motivi nazionalistici, non per motivi europei. Chiunque conosca la storia del rapporto tra la Francia e il Libano; chiunque conosca la storia della seconda guerra mondiale e sa che lì è nato il contrasto tra la Francia repubblicana e gli Stati Uniti, l'America

abbiamo sentito tutti i proclami contro il disarmo di Hezbollah, abbiamo ascoltato smentite anche clamorose della disponibilità al presidio del confine con la Siria. Sappiamo che vi sono rapporti dell'*intelligence* che continuano a dirci che di lì le armi stanno continuando a passare. Ma se il riarmo di Hezbollah andrà avanti (le intenzioni (le intenzioni cioè prevarranno sugli imprevisti della storia che noi in ogni caso ci auguriamo); se Israele tornerà a sentirsi minacciata della propria esistenza,

il dibattito che si è svolto in Aula sulla missione in Libano ha mostrato significative convergenze e legittime preoccupazioni. La domanda a cui siamo però chiamati a dare una risposta è fondamentalmente questa: la missione UNIFIL 2, e di conseguenza la partecipazione del nostro contingente, è utile all'obiettivo della pace in una regione così cruciale per la stabilità del Mediterraneo? Mediterraneo? Nel dibattito non ho sentito da parte di nessuno dei senatori intervenuti, nemmeno dei più critici tra loro, una risposta negativa a questa domanda. Del resto, la tregua che la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha ottenuto in Libano, tregua che tiene, è un risultato troppo prezioso per sottovalutarlo. E la missione UNIFIL 2 è parte integrante di quella risoluzione, le dà forza e credibilità. Allo stesso modo ho riscontrato nel dibattito una sostanziale concordanza su un punto di grande rilievo: e cioè che il nostro Paese, da tempo impegnato con efficacia in missioni internazionali di pace in tutto il mondo, ha il dovere e le capacità per essere in prima linea negli sforzi della comunità internazionale lì dove le sorti della pace vadano attivamente difese. Restano certo i rischi, che anzi sono destinati ad accrescersi a mano a mano che UNIFIL sarà chiamata a svolgere i suoi compiti per la rimozione delle cause del conflitto, oltre che per garantire la fine del conflitto. Nessuno ne è inconsapevole, meno che mai il Governo. I rischi sono certo relativi alla situazione sul terreno, alla presenza in Libano di una milizia pesantemente armata, ai motivi di dissidio tra Libano e Israele che permangono. Ma quei rischi discendono anche da un quadro internazionale più vasto. A nessuno sfugge che la guerra del Libano, pur innestandosi su cause storiche e locali, si è trasformata in una specie di frontiera avanzata di un conflitto potenzialmente più vasto. Né ci sfugge che un altro rischio, forse più immediato e imponderabile, si annida nella tattica da parassita della violenza che ha adottato Al Qaeda, che con estrema lucidità vede in ogni occasione di pace in Medio Oriente una minaccia mortale alla sua strategia di guerra totale. guerra totale. Se avessimo bisogno di una sola prova delle buone ragioni della missione in Libano, l'ostilità e le minacce di Al Qaeda al contingente di pace sono quella prova. Rischi quindi ci sono, e le preoccupazioni sono dunque giustificate. Ma questi rischi vanno contrastati in due modi, entrambi al centro dell'attenzione del Governo. Il primo è la chiarezza e la robustezza delle regole di ingaggio e su questo punto, anche relativamente al comportamento che i nostri soldati dovranno tenere nei confronti di miliziani armati o che traffichino in armi, il ministro Parisi ha dato informazioni, da me richiamate nella relazione introduttiva, che ci autorizzano a ritenere UNIFIL 2 più attrezzata e più pronta di UNIFIL 1 uno per svolgere i compiti che la risoluzione ONU le affida. I caschi blu non sono impotenti, senatrice Colli, non questa volta. Il secondo modo per contrastare i rischi di insuccesso della missione sta in un'evoluzione positiva della situazione internazionale, perché è evidente che solo nel quadro di un processo politico e diplomatico di progressiva distensione nell'area mediorientale la missione militare può ottenere risultati duraturi. L'uso della forza non può essere escluso nella ricerca della pace e su mandato delle organizzazioni internazionali, ma non può nemmeno essere auspicato come principale strumento di risoluzione delle controversie. Vorrei fare un'ultima osservazione rivolta a quei senatori che hanno messo in dubbio l'effettiva importanza di un voto *bipartisan* sulla missione in Libano. La sostanziale unità del Parlamento nel caso di missioni internazionali all'estero è un bene di estremo rilievo, non solo come espressione di sostegno e solidarietà nei confronti dei nostri soldati (essi sono effettivamente «eroi di pace», per usare l'espressione del collega Rotondi). Ma l'unità del Parlamento è cruciale anche, e vorrei dire soprattutto, per accrescere l'autorevolezza e il peso dell'Italia nelle scelte future della comunità internazionale, beni preziosi per l'interesse nazionale, chiunque sia al Governo. E questo vale più che mai nei prossimi due anni, in questo biennio in cui la nostra presenza nel Consiglio di sicurezza dell'ONU ci consentirà di esprimere una politica estera attiva e di farla pesare dove si decide, se ne saremo capaci. In questo momento, per ragioni non tutte dipendenti dalla nostra volontà o dalla nostra capacità, l'Italia è estremamente utile a ricostruire il tessuto di una politica unitaria della comunità internazionale, basata su una ritrovata *partnership* tra Stati Uniti ed Europa. Non indeboliamola per ragioni, seppur legittime, di contrapposizione politica, né per estenuare dibattiti che si riferiscono ad un passato che ha visto il Parlamento diviso, e sul quale ogni Gruppo parlamentare è pienamente legittimato a mantenere e a difendere il proprio convincimento. Stiamo per votare sulla missione in Libano, e su essa sola. Se il Senato è sostanzialmente d'accordo sulla sua necessità ed opportunità, lo dica con un voto ampio e forte. Il nostro voto non interromperà la dialettica politica, né impedirà a ciascuno di noi di esprimere liberamente la sua opinione, se e quando la situazione sul terreno o sulla scena internazionale dovesse cambiare. Per questo rinnovo il mio auspicio perché il Senato possa approvare ad ampia maggioranza il disegno di legge in esame. *(Applausi dei

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'Italia è stata eletta, praticamente all'unanimità, membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; ha avuto un ruolo decisivo per l'intervento in Libano, e presto avremo la guida del contingente internazionale in quel Paese. Siamo impegnati ad attuare la risoluzione 1701, una risoluzione *made* *in* *Italy*, così è stata definita dal senatore Tonini, perché nata dalla Conferenza di Roma che è stata la prima pietra verso il percorso che ha spento le fiamme in Libano. Abbiamo una concertazione molto stretta con la Germania, che il 1° gennaio assumerà la Presidenza dell'Unione Europea. Insieme a Spagna, Francia e Germania potremo esprimere nel Medio Oriente una politica ed una presenza dell'area dell'euro, che finalmente avrà un ruolo trainante.

un multilateralismo con i denti, come è stato definito dal senatore Polito, di un interventismo per la pace, di un pacifismo non isolazionista, come ha detto il senatore Tonini. Sono tornate le Nazioni Unite, la NATO, l'Unione Europea, e ringrazio il senatore Zanone per aver ricordato gli sforzi del nostro Governo per europeizzare la missione in Libano. Non vorrei guardare al passato, e tuttavia le Nazioni Unite, la NATO, l'Unione Europea ed il multilateralismo differenziano la situazione del Libano da quella dell'Iraq. Vorrei citare San Tommaso perché è stato citato dalla senatrice Brisca Menapace: bisogna distinguere frequentemente. Qui è proprio il caso di distinguere tra Iraq e Libano. Questi sono aspetti positivi di forma e di struttura che ci incoraggiano, e ci sono aspetti positivi sostanziali. Israele, per la prima volta nella sua storia, accetta la tutela internazionale e non si affida soltanto alle proprie forze, come ricordato dal senatore Polito. Gli Stati Uniti stessi sembrano essere passati dall'unilateralismo al multilateralismo;

l'europeismo di questo Governo è quello che punta ad un'Europa alleata degli Stati Uniti, ma un'alleata che sia autonoma, su un piano di parità, che convince e si fa convincere,

L'intervento in Libano, signori senatori, ha già prodotto il suo effetto; bisognerà vedere se sarà duraturo, ma un incendio è stato spento. Non si muore più e si discute sulla ricostruzione del Paese.

certo è che il prezzo del petrolio è sceso notevolmente e che per ogni 10 per cento di calo del prezzo del petrolio il nostro Paese risparmia quasi 3 miliardi di euro all'anno. In effetti, il petrolio, il gas, l'energia sono una componente importante nella crisi del Medio Oriente. Ringrazio la senatrice Pisa per essere sempre attenta a tale tema e per avercelo riproposto. L'incendio è stato spento, ma il fuoco cova tutto intorno. O lo si spegne dappertutto, o c'è il rischio che l'incendio divampi di nuovo. Altro che trionfalismo. Certo, la situazione richiede un intervento lungo, pericoloso e difficile. Il Libano non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Deve essere l'inizio di una pacificazione più generale. Il Libano è il primo cerchio, la pace parte da lì:bisogna rafforzare il Governo Siniora e pacificare due Stati sovrani, Israele e Libano. Lo ha ricordato il relatore Polito ed è un particolare non da poco: Bisogna ottenere il rilascio dei soldati israeliani rapiti, affrontare il tema delle fattorie di Shebaa occupate dal 1967 - come si sa - da Israele. a quel momento erano parte del Golan siriano, mentre oggi tutti accettano che siano libanesi. Sono un alibi e una giustificazione (ciascuno la può pensare come crede) per il fatto che Hezbollah sia restato in armi.

Il Libano è il primo cerchio ma - come si ricordava poco fa - la crisi palestinese è la madre di tutte le crisi, l'alibi - anche qui - o la giustificazione di tutte le violenze. So bene che il terrorismo islamico non morirebbe anche se si risolvesse il problema palestinese. Ciò nondimeno, risolvere il problema palestinese è condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la pace in Medio Oriente, nel Mediterraneo e nel mondo. affrontare subito la crisi perché il tempo non gioca a nostro favore. Bisogna prendere per le corna la questione palestinese. Tutto si tiene. Gli attori in Medio Oriente sono tanti. Bisogna coinvolgere anche la Siria e l'Iran. Ha fatto bene il senatore De Gregorio, presidente della Commissione difesa, a ricordarlo nel suo intervento: sarebbe un errore escludere l'Iran, a meno che esso non si escluda da solo. Il primo cerchio è il Libano, il secondo la Palestina e il terzo sono il Golan, l'Iran, con la sua questione nucleare irrisolta, e l'Iraq. Tutto si tiene. Ad esempio, è impossibile stabilizzare l'Iraq senza che Teheran sia coinvolta. È impossibile trovare un *modus* *vivendi* con Teheran senza risolvere la questione palestinese e senza arrivare a una pace stabile che trovi il consenso anche di Hezbollah e di Hamas e viceversa. Tutto si tiene e anche l'Afghanistan, dove la NATO ha svolto un intervento di emergenza. Ma, finita l'emergenza, la NATO deve essere sempre più affiancata dalla comunità internazionale, che deve preoccuparsi dell'incendio afgano come di quello mediorientale. A proposito di Afghanistan, vorrei soltanto dire questo: lì non siamo come volonterosi, non siamo come siamo stati in Iraq: siamo all'interno di una comunità, all'interno di una alleanza, e quando si è all'interno di una comunità e di una alleanza non sono possibili scelte unilaterali. A febbraio, un generale italiano guiderà in Libano spagnoli, francesi e tedeschi. È possibile dire, nel contempo, agli spagnoli, ai francesi e ai tedeschi «vi guidiamo in Libano, ma in Afghanistan ce ne andiamo e vi lasciamo da soli»? Non credo. Saremmo, in questo caso, non al multilateralismo, ma all'isolamento, non alla solidarietà europea, ma alla divisione dell'Europa. Le ragioni di chi sostiene che in Afghanistan la situazione richiede una iniziativa, tuttavia, sono ragioni che vanno ascoltate con attenzione e rispetto, perché sono fondate: le critiche vanno sottolineate e se ne deve tenere conto. Ad esempio, c'è una contraddizione che è sotto gli occhi di tutti: la comunità internazionale presidia l'Afghanistan, lavora al *nation-building* dell'Afghanistan; nel contempo, l'Afghanistan è diventato un narco-Stato: il primo fornitore al mondo di eroina, infetta il mondo fornendo il 90 per cento della produzione di oppio. L'opposizione, signori senatori, si accinge dunque a votare questo provvedimento. A parte la Lega, il senatore Guzzanti, la senatrice Colli, forse il senatore Selva che hanno espresso forti riserve, ringrazio l'opposizione per questo voto e per questo consenso. D'altronde, mai una missione ha avuto un appoggio più ampio: è d'accordo Israele ed è d'accordo ed è presente militarmente il Paese che ospita Al Jazeera, Al Jazeera, il Qatar; sono d'accordo gli Stati uniti e la Cina, che pure partecipa alla missione; soprattutto, sono d'accordo in Europa la destra e la sinistra: è d'accordo la sinistra che governa la Spagna e la destra che governa la Francia e, in Germania, la sinistra e la destra che governano insieme. L'occasione di unità che viene da Libano a livello mondiale è una occasione di unità anche per il nostro Parlamento. Sento, naturalmente, negli interventi dell'opposizione una costante critica, un allarme continuamente ripetuto, anche da chi si accinge a votare a favore nell'opposizione stessa: riguarda gli Hezbollah e il loro disarmo. Vorrei essere chiaro su questo punto: non siamo in Libano per combattere contro qualcuno, non scommettiamo sulla guerra civile del Libano, ma sulla pacificazione del Libano. Scommettiamo perciò sulla possibilità che lo Stato sovrano libanese si rafforzi. Hezbollah è un movimento politico e militare al tempo stesso: contiamo che il politico assorba il militare e non l'opposto. Vale l'osservazione fatta dal ministro degli esteri D'Alema in Commissione esteri, già ricordata dal senatore Polito: l'impianto della risoluzione delle Nazioni Unite è che il disarmo di Hezbollah sia il risultato dell'azione politica e militare del Governo libanese stesso, assistito dalla comunità internazionale e dall'UNIFIL. Ciò evidentemente significa che la forza UNIFIL non ha il mandato di disarmare direttamente Hezbollah, ma ha il mandato di contribuire a rendere possibile questo risultato. Infine, e concludo, signori senatori, un'osservazione più generale che riguarda tutte le missioni e non solo quella del Libano: stabilità, certezze, certezze che durino non sei mesi, ma quanto l'esercizio finanziario, ovvero un anno sono obiettivi da raggiungere. Per questo avevamo presentato, come Governo, l'articolo 188 della finanziaria. Si è avanzato il timore che la finanziaria fosse una sede impropria per affrontare e risolvere questo problema di stabilità, si è temuto che potesse essere impedito un dibattito politico pieno su tutte le missioni militari. Maquesta mattina, in Commissione esteri, si è raggiunto un utile punto di equilibrio: con un voto unanime dell'intera maggioranza e dell'intera opposizione, è stato conservato il solo primo comma dell'articolo 188, il che dà stabilità e certezza, perché fissa per tutto l'anno lo stanziamento al mantenimento delle nostre truppe all'estero; un decreto, con decorrenza 1° gennaio, autorizzerà poi tutte le singole missioni, ma le autorizzerà non per sei mesi, bensì per un anno, il che non impedirà certo - e il Governo è pienamente d'accordo - un costante controllo e monitoraggio del Parlamento. Questo problema poteva creare divisioni nella maggioranza. Non lo ha creato perché si sono contemperate due esigenze: da una parte consenso e controllo del Parlamento; dall'altra, stabilità e certezze anno per anno e non semestralmente per le nostre missioni, secondo i ritmi, quindi, dell'esercizio finanziario e non secondo i ritmi della precarietà. Ringrazio ancora il Senato per il voto quasi unanime che si accinge ad esprimere. Voti come questo indicano che l'Italia, come tutte le grandi nazioni, sa individuare il proprio interesse nazionale e sa renderlo ampiamente condiviso.

Il G1 esprime apprezzamento per le nostre Forze armate impegnate in tutte le missioni internazionali di pace in corso, nel rispetto dei valori espressi dall'articolo 11 della Costituzione, e impegna il Governo a sostenerne l'operato.

Il Governo condivide il parere espresso dal relatore ed

esprimiamo, come detto in modo molto chiaro dall'ordine del giorno, apprezzamento per il ruolo delle nostre Forze armate impegnate nelle missioni internazionali di pace. Tuttavia vogliamo segnalare all'Assemblea, perché rimanga nel Resoconto, che riteniamo assolutamente strumentale che si cerchi, attraverso un ordine del giorno, di determinare una continuità fra tutte le missioni internazionali. Ciò riteniamo sia un falso sia storico che politico, non solo perché sulla vicenda dell'Iraq avevamo espresso differenti valutazioni e votazioni; non solo perché sulla vicenda dell'Iraq questa maggioranza ed il Governo hanno deciso conseguentemente rispetto alle proposte fatte in campagna elettorale; non solo perché per quanto riguarda l'Afghanistan abbiamo sempre votato in modo contrario; non solo perché per l'Afghanistan riteniamo necessaria un'azione politica di fuoriuscita da quella situazione pericolosa per il nostro Paese. Soprattutto, signor Presidente, vogliamo sia evidenziato nella nostra discussione il fatto che c'è invece una discontinuità reale e politica nella politica internazionale che il nostro Governo ha adottato in questi ultimi mesi. Mi riferisco al nuovo ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, in particolare nel rapporto con il mondo arabo, e ad una politica di pacificazione in Libano che deve arrivare a costruire le condizioni per giungere ad una pace vera tra

multilateralismo; al ruolo diverso rispetto all'ONU che riprende iniziativa e capacità di intervento nelle crisi internazionali; al rapporto vero non di sudditanza con gli Stati Uniti, un rapporto per cui, dentro una vera alleanza, ci si confronta alla pari. Credo che questi siano elementi decisivi di discontinuità, che non possono essere negati. Per tali motivi, Presidente, riteniamo sia assolutamente strumentale utilizzare un ordine del giorno per rivendicare una continuità che invece non c'è. *(Applausi STORACE *(AN)*. L'intervento che mi ha preceduto ci solleva quanto a responsabilità, perché consente di fare chiarezza e di poter raggiungere l'obiettivo di un voto largamente maggioritario per la missione in Libano anche con il nostro concorso. Vede, Presidente, vede, Ministro, se non avessimo presentato un ordine del giorno identico a quello del relatori, ovvero se quest'Aula si fosse accontentata del semplice scambio di opinioni tra relatore e Governo, oggi non sarebbe venuto allo scoperto quello che abbiamo sentito poc'anzi. A parti invertite, con la nostra maggioranza di allora, questa missione sarebbe partita; con le parti attualmente in campo, con voi al Governo e noi all'opposizione,

non si farebbe un pezzo di strada in avanti. Vorrei dire all'autorevole rappresentante della sinistra radicale - che almeno ha detto le cose in cui crede, senza fingere in questo caso - che il testo di questo ordine del giorno ribadisce quello che è scritto nella Costituzione, ribadisce che le missioni che sono partite per volontà dei Governi della Repubblica hanno avuto il sigillo dei Capi dello Stato, a cominciare dal presidente della Repubblica Ciampi, in omaggio all'articolo 11 della Costituzione. Alla Camera non è stato fatto votare quel documento, qui viene fatto votare ed è bene che si smantelli l'ipocrisia che c'era attorno a tale questione. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione Comunista si asterrà dal votare questo ordine del giorno.

oggi il collega senatore Storace scopra che veniamo allo scoperto. Noi allo scoperto ci siamo sempre stati, nella nostra linea pacifista e riteniamo, anzi, che questo ordine del giorno abbia

«L'Italia ripudia la guerra». Noi riteniamo che alcune delle missioni in cui sono impegnate le Forze armate italiane non siano missioni di pace, di pacificazione e di ricostruzione civile ma siano... È inutile che fate gazzarra. Ne abbiamo discusso mille volte, non ci spaventiamo certo se levate degli ululati. Se vogliamo discutere, discutiamo, in un confronto serio. Riteniamo

la missione militare in Iraq, a Nasiriya (che non a caso questo Governo e questo Parlamento hanno ritirato), non siano equivalenti alla missione in Afghanistan, a cui pure siamo contrari e che abbiamo votato all'interno della coalizione

anche sulla annosa questione della pace fra Israele e Palestina, con la costruzione dello Stato palestinese e la garantita sicurezza lo Stato d'Israele. Di questo stiamo parlando. Allora, strumentalismi, politicismi, cosiddette trappole, i «venuti allo scoperto» sono parole senza senso. Stiamo parlando di vite umane, di pace e di guerra. Il nostro apprezzamento per i soldati italiani

La Lega, Presidente, non potrà votare questo l'ordine del giorno, anche perché

dice sì a tale missione lo fa con mille, se non mille e uno, retropensieri. Infatti, al di là di fingere di allinearsi con la risoluzione ONU 1701, di fatto si pensa già non tanto a disarmare i terroristi, ma sulla falsariga delle richieste del Governo regolare libanese a tutte le forze presenti sugli scenari di guerra di aiutare a migliorare e modernizzare l'esercito, il fornire armi all'esercito regolare non farà altro che finire per riarmare effettivamente Hezbollah e i terroristi e punire Israele, che si troverà imbrigliato

L'elogio della sincerità è un complimento, non è una mancanza di riguardo, perché si svelano le ragioni profonde che militano quando non vi è l'obbligo di credere e obbedire senza combattere. Questa mi pare sia la realtà. *(Applausi dal che c'è l'opposizione democratica, la quale, per un valore superiore, che non è di parte, ma riguarda la pace nel mondo, in quel settore particolare, dove sono impegnati nostri soldati, fa il gesto che voi non avete fatto con noi. In quello sta la distinzione, perché voi offendete il Presidente della Repubblica, che vota per voi,

c'è la pace e se si combatte per la pace e la democrazia dovremmo teoricamente, in politica estera, essere tutti dalla stessa parte. Capisco che voi non riusciate ad uscire dalla vostra parte salvo quando siete costretti dal voto di fiducia che vi impone la mordacchia per la quale non fate il vostro dovere di coscienza.

ringrazio per avermi dato la parola, seppure alla fine.

PISANU *(FI)*. Rispetterò la sua esortazione alla brevità, signor Presidente. A me sembra singolare la motivazione

cosa che mi sembrerebbe estremamente pericolosa e in netto contrasto con le affermazioni fatte anche recentemente

che sono state fatte nei giorni scorsi quando eravamo in campagna elettorale in cerca di voti alle Nazioni Unite per la candidatura per la votazione dell'ordine del giorno G9 perché manteniamo fermo e alto il richiamo ai tre pilastri della politica estera italiana. Chi li vuole negare li neghi con il voto!

del Ministro degli affari esteri. Evidentemente il ministro D'Alema la pensa in modo diverso da noi. È chiaro che la contrarietà da parte del Governo è relativa all'ultima parte dell'ordine del giorno laddove si afferma «con la tradizionale coessenzialità dei tre pilastri fondamentali della politica estera italiana quali l'ONU,

l'ordine del giorno G7 testé approvato non ha le caratteristiche di una trappola, né surrettiziamente vuole introdurre giudizi politici sulle missioni internazionali del passato,

nel complesso e con grande ampiezza di considerazioni la Commissione esteri e la Commissione difesa. Ci era sembrato giusto recuperare lo spirito di un ordine del giorno analogo, che era stato presentato alla Camera e che aveva visto il consenso del Governo. L'ordine del giorno G9, invece, introduce - questo sì, surrettiziamente - valutazioni politiche sul senso e sul significato delle altre missioni; quindi, rompe quella

vorrei ricordare che il ministro degli affari esteri D'Alema è da ieri impegnato in Lussemburgo al Consiglio e quindi non ha potuto essere presente per tale motivo. D'altronde, si è saputo soltanto questa mattina che il Senato avrebbe concluso i suoi lavori sul Libano in giornata. Vorrei aggiungere qualche parola sulla questione dell'ordine del giorno G9. In questo ordine del giorno si sottolinea che esistono tre pilastri tradizionali, sempre seguiti dalla politica estera italiana: l'ONU, la NATO e l'Unione Europea. Il Governo è dell'opinione che non ci sia stata continuità nel sostenere questi tre tradizionali pilastri, perché tale tradizione è stata in qualche modo spezzata proprio dalla vicenda irachena, in cui non c'erano tre pilastri, ma forse mezzo. Intendo dire che in Iraq non c'era la NATO, non c'era l'Unione Europea e c'era a metà il sostegno delle Nazioni Unite. Presidente, onorevoli senatori, era apparso chiaro nella discussione svolta nelle Commissioni esteri e difesa che ci fosse una condivisione di intenti sul voto dell'ordine del giorno G1. In In Aula prendiamo atto che ci sono posizioni diversificate, a differenza di quanto avevamo immaginato nella discussione all'interno delle Commissioni. L'atmosfera di condivisione ovviamente porta a delle conseguenze chiare; io stesso mi sarei permesso di chiedere al collega Schifani e agli altri firmatari dell'ordine del giorno G9 di ritenersi soddisfatti dell'approvazione collettiva dell'ordine del giorno G1, che dava atto della continuità delle nostre missioni di pace, alla quale teniamo, perché quando si tende la mano

giorno G9, perché i distinguo, se devono esserci, vanno bene da una parte e dall'altra, anche se rovinano qualche volta l'atmosfera di condivisione con la quale ci auguravamo di arrivare al voto questa sera. Presidente, signor Vice ministro, onorevoli relatori, avrei piacere che fossero evidenti in quest'Aula le cose sulle quali siamo d'accordo, che sono molto importanti e numerose. Il disaccordo, non è una sorpresa, può riguardare talune parti della conduzione della politica estera italiana. Per quanto riguarda le cose sulle quali siamo d'accordo, a nome dell'UDC che voteremo a favore della conversione del decreto-legge sulla missione in Libano. Non è per niente un fatto scontato e ovvio. Siamo d'accordo perché riteniamo che questa missione militare di pace sia nel solco dell'articolo 11 della Costituzione. Abbiamo ritenuto e riteniamo che tutte le missioni italiane all'estero siano nel solco dell'articolo 11 della Costituzione, ossia siano missioni di pace. Tali le ha ritenute la Camera dei deputati, che si è espressa a favore di questa interpretazione.

Costituzione». Sono due punti fondamentali di intesa larghissima: la missione in Libano ci vede concordi e le missioni in corso sono tutte nel solco dell'articolo 11 della Costituzione. quale parte l'ordine del giorno G9 dice cose che alcuni ritengono impropriamente affermate? Siccome sono uno dei firmatari dell'ordine del giorno, vorrei che fosse chiaro che noi stiamo sostenendo, d'accordo con tutti i Gruppi presenti in Senato (abbiamo votato l'ordine del giorno G1 e voteremo la missione in Libano), e stiamo affermando che la politica estera italiana non è in aggiunta all'articolo 11 della Costituzione (lo dico ai colleghi Capigruppo e a tutti i colleghi senatori degli altri Gruppi). Noi non diciamo, nell'ordine del giorno G9, che vi è l'articolo 11 della Costituzione, in base al quale sono previste le missioni in corso, e vi sono i princìpi e i pilastri della politica estera, che sono altra cosa. Diciamo, dal punto di vista letterale (occorre capire!), che sono in linea con l'articolo 11 della Costituzione e «pertanto» con la tradizionale politica estera italiana. Quel «pertanto» è rafforzativo dell'articolo 11 della Costituzione, non è oppositivo. Ecco perché il nostro ordine del giorno, in qualche modo, politicamente è riassunto dall'ordine del giorno G1 e contiene una specificazione che può sorprendere che rappresenti motivo di divisione. Non stiamo sostenendo che vi è il principio di pace della Costituzione e vi sono le alleanze internazionali dell'Italia, sulle quali vi può essere dissenso. Ecco perché io insisto e chiedo al vice ministro Intini e ai colleghi relatori di riflettere ancora una volta su questo fatto vi è una politica estera basata sull'articolo 11 della Costituzione e «pertanto», non in alternativa o in aggiunta, vi sono vi sono questi temi di politica estera, che possono essere visti in modo diverso dai diversi Governi della Repubblica. Non c'è niente di scandaloso che vi possa essere un Governo che accentui di più l'Unione Europea e un po' meno la NATO e un altro che accentui di più la NATO e un po' meno le Nazioni Unite; non c'è nulla di sconvolgente, purché si capisca che dentro questo recinto ci siamo tutti (come ci siamo tutti). Ribadisco che il Gruppo UDC vuole sottolineare le ragioni dell'intesa sulle quali quest'Aula si pronuncia, molto più delle non facilmente comprensibili ragioni di divisione, che se riguardano singoli Governi sono del tutto legittime, ma che non possono riguardare atti decisivi di politica estera. Per queste ragioni, chiedere che il Governo ragioni sull'ordine del giorno G9; qualora il Governo lo accogliesse, noi non insisteremmo per la votazione.

poi al riguardo, nella mia dichiarazione di voto, in termini più espliciti e più compiuti la nostra posizione.

nella parte finale, fa riferimento all'ONU, alla NATO e all'Unione Europea. C'è una parte di queste missioni, nella quale non c'è la NATO e non c'è l'Unione Europea e l'ONU è intervenuta soltanto in una seconda fase. fase. Per tali ragioni credo che questa definizione letterale sia più restrittiva e limitativa rispetto alla prima che abbiamo già approvato.

Signor Presidente, una questione che continueremo a far fatica a comprendere è perché si continui a voler nascondere la verità. Il vice ministro Intini, riferendosi alla missione irachena, ha persino detto che non si sarebbe nemmeno retta su mezzo pilastro. Non capiamo perché ci si ostini a mantenere queste posizioni anche in un dibattito serio, sereno, dove la maggioranza e l'opposizione sono arrivate a condividere alcune posizioni. Anche la missione irachena è stata giustificata sulla base di risoluzioni ONU. Il precedente Presidente della Repubblica aveva dato il pieno assenso all'intervento italiano a conflitto terminato.

europei presenti, con tre (Germania, Grecia e Gran Bretagna) impegnati soltanto in supporti navali. Non possiamo continuare a raccontare bugie, perché a noi sembra che le missioni vengono supportate o meno in base al tasso di maggioranza che corre nel sangue al momento in cui si fanno. Queste cose non ci piacciono!

Presidente, credo che sia giusto fare una distinzione molto netta tra due livelli del nostro dibattito e del nostro confronto. Siamo in una fase delicata; stiamo per dare il via libera ad una missione rischiosa e doverosa, come abbiamo detto nel dibattito di questa mattina. Credo non ci debbano essere tra di noi trucchi o trappole. Ci sono due livelli diversi del nostro discorso; uno è il livello della legittimità delle missioni, l'altro è il livello del dibattito politico. Sulla legittimità credo che sia stato un errore da parte di alcuni colleghi della maggioranza - come per altro da parte dei colleghi della Lega - non votare l'ordine del giorno G1, perché credo che non ci possano essere dubbi sul fatto che la legittimità ex articolo 11 della Costituzione sia sempre stata rispettata. Altra cosa però è voler riscrivere la storia nell'Aula del Parlamento. Si è detto che non si deve riscrivere la storia nelle aule dei tribunali, ma non si può riscrivere la storia nemmeno nelle Aule del Parlamento. Sull'opportunità - che è altra cosa dalla legittimità - della missione in Iraq questo Parlamento si è diviso. Non ha senso, non ha senso, non è intellettualmente onesto - vorrei dire ai colleghi dell'opposizione - in questo momento voler riscrivere surrettiziamente questa storia. Sulla legittimità possiamo essere uniti, sull'opportunità politica siamo divisi e questa divisione è bene che resti perché fa parte della nostra storia; dobbiamo accettarla con serenità, non usarla gli uni contro gli altri, ma è un'operazione non seria quella di pensare che si possa passar sopra a questa diversità con un ordine del giorno.

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi alle ore 18, in relazione all'andamento dei lavori della 2a Commissione permanente e per consentire alla medesima di concludere nei tempi stabiliti l'esame in sede referente del decreto‑legge in materia di intercettazioni telefoniche, ha deciso che l'Assemblea tornerà a riunirsi domani mattina alle ore 11,30, nel presupposto della conclusione del provvedimento da parte della Commissione. Domani mattina, fino alle ore 11,30, potranno pertanto riunirsi anche le altre Commissioni permanenti, con particolare riguardo ai provvedimenti previsti dal calendario. **Ripresa della discussione dei esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, nel presupposto che le norme contenute nel provvedimento rientrino nelle fattispecie richiamate dal comma 4, dell'articolo 1, della legge finanziaria n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) in materia di interventi imprevisti e straordinari a tutela della sicurezza del Paese e osservando quanto segue: - in relazione all'articolo 9, contenente la copertura finanziaria del provvedimento, si prende atto che il Governo ha affermato che maggiori entrate per 400 milioni di euro sono state accertate sul capitolo 1033/1 (imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni), si ribadisce l'urgenza di acquisire l'atto amministrativo necessario per accertarne formalmente l'esistenza ed inglobare nel bilancio la cifra in questione;» una copertura sulla parola - - «in relazione all'articolo 6-*bis*, il parere è di nulla osta nel presupposto che, come dichiarato dal Governo, non sussistono ipotesi di richieste emulative da parte di altri corpi non facenti parte dell'Esercito».

Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare l'emendamento 10.100, lasciando al collega Divina l'incombenza di illustrare L'articolo 10 del decreto in esame fa riferimento a non meglio precisati rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare UNIFIL *plus*.

Senatrice Finocchiaro e senatore Iannuzzi, Da qui sembra suonato l'intervallo! Il Senato è aperto e sta lavorando. *(Applausi

Senatore Manzella, mi rispedisce a posto il senatore Iannuzzi che sta importunando tutti i colleghi? La ringrazio. Prego, collega Stiffoni, *(LNP)*. Non sono noti i criteri oggettivi che regolano l'erogazione di rimborsi concessi dalle Nazioni Unite ai Paesi che mettono a disposizione le proprie truppe per l'effettuazione degli interventi militari internazionali deliberati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

STIFFONI *(LNP)*. È ignota anche l'entità dei rimborsi che riceverà la Francia, Paese che contribuisce all'UNIFIL *plus* con un contingente di entità inferiore a quello offerto dall'Italia.

merito all'esatto ammontare delle risorse che le Nazioni Unite corrisponderanno all'Italia e alla Francia, a parziale ristoro delle spese che saranno sostenute per la partecipazione di militari italiani e francesi alla missione, nonché i tempi prevedibili in cui saranno effettivamente erogati al nostro Paese. Infatti, signor Vice Ministro, mi risulta che il rimborso che la Francia ha ottenuto, solo per essere stato gradevolmente richiesto, sia molto superiore a quello che l'ONU darà all'Italia.

di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti». Vorrei aprire e chiudere una parentesi: non è specificato che tale ripristino di scorte e manutenzione si riferisca soltanto ai materiali usati dalle nostre Forze armate. Forse ve lo siete dimenticato. In ogni caso, con l'emendamento 10.100 noi della Lega Nord desidereremmo che i rimborsi fossero destinati

vorrebbe che fosse modificato l'articolo 5 del decreto-legge e che ai nostri militari non fosse applicato il codice penale militare di pace, ma il codice penale militare di guerra. Le motivazioni sono semplici, signor Presidente: noi non sappiamo (ma non è questo il problema) e i nostri militari in Libano non sanno quale atteggiamento dovranno tenere nel caso in cui le nostre Forze armate fossero attaccate da Hezbollah, da Israele, oppure da entrambi, o ancora nel caso in cui entrambi riprendessero le ostilità. Non è stato scritto e non è stato previsto, Presidente, per esempio, l'immediato ritiro delle nostre truppe, qualora tra Hezbollah e Israele il conflitto precipitasse e le ostilità riprendessero.

Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo per pronunciare il nostro voto su un disegno di legge utile a convertire il decreto-legge 28 agosto scorso, concernente la partecipazione italiana alla missione UNIFIL in Libano. La missione in questione, come è ben noto, opera attraverso un mandato stabilito dalla risoluzione 1701 dell'ONU, il cui impianto vuole che il disarmo di Hezbollah sia il risultato dell'azione politica e militare del Governo libanese stesso, assistito dalla comunità internazionale e dall'UNIFIL. L'UNIFIL dunque, è bene sottolinearlo, è una forza di interposizione, neutrale rispetto alle parti in conflitto, che comandata sul campo proprio dalle nostre truppe ha ottenuto da subito il significativo effetto di un «cessate il fuoco» permanente, dando uno *stop* alla spirale di stragi che si era innescata nell'area israelo-libanese. L'Italia ha giocato e gioca, quindi, un ruolo fondamentale per la conduzione ed il prosieguo di tale missione, avendo dimostrato già autorevolezza e credibilità della sua posizione sin dal 18 agosto; giorno in cui, insieme agli altri colleghi delle Commissioni esteri e difesa, ci siamo ritrovati in Parlamento per dare un convinto sostegno alla missione tramite una risoluzione votata, quando ancora aleggiavano incertezze forti negli altri Paesi europei. Quello del 18 agosto è stato l'ottimo inizio di un percorso che deve necessariamente proseguire con la rapida conversione del decreto al nostro esame, con cui il Governo ha disposto interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano ed il rafforzamento del contingente militare e la missione UNIFIL 2; decreto approvato dalla Camera con modificazioni relative agli oneri finanziari. La missione UNIFIL certamente si prospetta ancora lunga ed impegnativa poiché tanti ancora sono i compiti che i nostri militari dovranno portare a termine. Solo per ricordarne alcuni, i nostri 1.500 militari già schierati in Libano, a cui se ne affiancheranno altrettanti nei prossimi mesi, sorvegliano costantemente, senza mai abbassare la guardia, sulla cessazione delle ostilità; affiancano le forze libanesi perché queste possano disarmare Hezbollah. Non dimentichiamo a tale proposito che tale obiettivo deve essere conseguito dall'azione politica e militare del Governo libanese stesso, che ha bisogno di riaffermare la propria sovranità statuale troppo spesso messa in discussione dalle milizie armate di questa o di quella formazione politica o etnico-religiosa esistente al suo interno, al fine di riacquistare credibilità anche sul piano internazionale. Ancora, il nostro esercito è impegnato a sostenere e controllare l'embargo al traffico di armi ed a contribuire al ristabilimento delle condizioni normali di vita delle popolazioni civili, che hanno subìto tante devastazioni e sofferenze. A tal proposito, voglio esprimere un sentito ringraziamento a quanti prestano tutti i giorni in condizioni altamente rischiose la propria grande esperienza e professionalità. Concludendo, vogliamo augurarci che il nostro impegno attivo in Libano possa ricevere, con la votazione odierna, il più ampio sostegno possibile poiché all'articolo 11 della nostra Costituzione detta, quale compito fondamentale della nostra nazione, quello di adoperarsi per il raggiungimento di un ordine internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli. L'Italia ha dunque l'obbligo di contribuire affinché si ristabilisca in modo efficace e duraturo la pace nelle terre del Libano e negli Stati confinanti del Medio Oriente, anche per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa stessa. Ecco perché dichiaro, a nome del Gruppo che rappresento Popolari-Udeur, il voto favorevole ed essendo vicepresidente del Gruppo Misto,

Lo facciamo convintamente e responsabilmente, consci che questa scelta corrisponda all'interesse strategico dell'Italia. La stabilizzazione del Medio Oriente è, infatti, elemento dirimente nel processo per promuovere e favorire il superamento di tensioni tra mondo occidentale e mondo musulmano; unico vero antidoto alla lotta contro il terrorismo e di conseguenza primario interesse per il nostro Paese. Altrettanto fondamentale è che il nostro Paese rispetti gli impegni assunti a livello internazionale, disattendere i quali provocherebbe una grave perdita di credibilità e di prestigio internazionale. Altri due elementi ci spingono a votare a favore: da una parte la perfetta coincidenza e quindi la continuità della politica estera del Governo Berlusconi e dall'altra il dovere morale di cercare, anche a livello parlamentare, di dare il massimo sostegno alle nostre Forze armate impegnate in una missione così delicata e rischiosa. Per inciso, che la politica estera così interpretata dia i suoi frutti è dimostrato dal risultato plebiscitario con il quale ieri l'Italia è stata eletta all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, come molti osservatori internazionali hanno evidenziato, il nostro impegno in numerose missioni di pace sotto l'egida dell'ONU ha avuto un peso rilevante. La mia dichiarazione di voto potrebbe finire qua, se non ci fossero alcuni aspetti critici che ritengo giusto analizzare. In particolare vorrei porre l'attenzione sull'atteggiamento di molti colleghi della maggioranza, per fortuna non tutti. Non vedo più il relatore e vedo che il Governo è praticamente assente: evidentemente questa è l'attenzione con la quale il Governo e il relatore di maggioranza si prestano In particolare, dicevo, vorrei porre l'attenzione sull' atteggiamento che molti colleghi della maggioranza hanno tenuto: anziché ricercare, su questioni di tale rilievo, il più ampio consenso possibile, hanno fatto a gara con le loro dichiarazioni per marcare una discontinuità con la politica estera del Governo precedente. Lo ha detto con chiarezza il relatore nella sua replica: è un bene per tutto il Paese che ci sia un largo consenso parlamentare, lo sforzo dobbiamo farlo tutti, ma vedo che la maggioranza predica bene e razzola, come al solito, nella maniera che le è più consona. Non credo quindi che l'atteggiamento tenuto da grande parte della maggioranza corrisponda all'interesse generale. Credo piuttosto che sia legato al maldestro tentativo di imporre ai propri compagni il «contrordine»; dopo avere agitato le piazze con manifestazioni, maree, girotondi, bandiere arcobaleno dappertutto, giuramenti solenni per sostenere: «Mai più guerra, mai più interventi armati, senza se e senza ma!», oggi bisogna rimangiarsi tutto. E quindi occorre dire «Sì» alla più vasta ed importante missione militare del nostro Paese, ma come ricordato da qualche collega dell'opposizione basta chiamarla «aiuto alla cooperazione», dire che è in discontinuità con il Governo Berlusconi, così la coscienza è tranquilla e quindi si può procedere. Comunque, prendiamo atto con soddisfazione che anche in questa circostanza vi siete ravveduti e avete cambiato idea. Peraltro non è la prima volta e anzi vi succede con una certa frequenza: oggi rispetto al passato siete i paladini del libero mercato, delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni, sostenete l'Unione Europea, anzi secondo voi siete gli unici ad avere il dogma dell'europeismo, sostenete la Nato, prendete le distanze dal comunismo dell'Unione sovietica, dai fatti di Ungheria e di Cecoslovacchia, insomma siete colpiti da quello che il vice ministro Visco chiamerebbe il «ravvedimento operoso». Di questi vostri ravvedimenti siamo soddisfatti, anche se gradiremmo che la volta prossima, quando vorrete ancora indicarci la via del bene, voi che avete verità in tasca, lo spiegaste forse con un po' meno saccente sicumera e con più Per quel che riguarda questa vicenda e per conoscere le vere ragioni del vostro cambiamento credo che a questo punto non si possa fare altro che attendere il secondo atto di un libro ormai diventato famoso, che non sarà «La missione UNIFIL 2», ma «La grande bugia 2». del tutto evidente che avremo la possibilità di scoprire quando e perché dimostrerete di aver cambiato, anche in questa circostanza, atteggiamento. Per quel che ci riguarda, per il bene che vogliamo al nostro Paese, per il senso di responsabilità nei confronti dei nostri uomini impegnati in quel fronte, nonostante i vostri atteggiamenti, nonostante la discutibile dimensione della missione

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'invio del contingente italiano nel Libano del sud nella missione UNIFIL, in seguito alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rappresenta sicuramente un positivo ritorno dell'Italia sullo scacchiere mediterraneo per una missione di pace. É prima di tutto da segnalare il carattere universalmente condiviso della necessità di una forza di interposizione che separi l'IDF, l'esercito israeliano, dalle zone controllate dalle milizie Hezbollah. È raro trovare simile unanimità rispetto all'invio di una forza armata. L'unanimità del sentimento mondiale rispetto all'invio è senz'altro dovuto al fatto che non possono sussistere dubbi sulla natura della missione che è veramente di pace. Non si tratta quindi di azione percepita come offensiva o al servizio di interessi diversi da quelli proclamati. Il fine è quello di interrompere i criminali lanci di razzi sulla popolazione israeliana e le conseguenti forse sproporzionate rappresaglie di Tsahal. Di questa necessità sono coscienti entrambe le parti belligeranti che hanno quindi salutato con favore la notizia dell'invio del contingente italiano, un fatto fondamentale, l'accordo delle parti. Separando i belligeranti, controllando i confini, assicurando la pace il contingente italiano consentirà che il Libano possa ricostruirsi liberamente nel pieno esercizio del suo diritto di autodeterminazione. qualcosa di indispensabile per il Paese dei cedri, passato dallo *status* di gemma del Medio Oriente a territorio oggetto di feroce scontri tribali e religiosi, nonché terreno di scontro tra altri Stati e che sia l'Italia a favorirlo deve essere per il nostro Paese motivo di legittima fierezza. Proprio il riconoscimento del suo ruolo ha permesso all'Italia di esercitare fin d'ora il comando strategico della forza UNIFIL presso il Dipartimento ONU per il *peacekeeping* e di ereditare dalla Francia quello delle forze sul terreno dal febbraio 2007. Siamo di fronte nuovamente ad un elemento altamente positivo che premia la professionalità delle nostre Forze armate, che peraltro già nel 1982 avevano dato in Libano ottima prova delle loro capacità al comando del generale Angioni. Professionalità e accettazione da parte della popolazione, che valsero ai nostri soldati di non conoscere i tremendi attacchi suicidi che subirono invece i *marines* e i parà francesi, sono state tali da indurre anche gli Stati Uniti a insistere perché l'Italia intervenisse un quarto di secolo dopo. La missione UNIFIL con comando italiano dimostra che gli europei sono perfettamente in grado di schierare contingenti, che in effetti la legittimità internazionale per loro è un valore e che gli interventi devono avere per obiettivo solo il ripristino della pace. Se gli europei sono oggi in grado di affermare in positivo un'identità anche militare che non inclina la solidarietà transatlantica è anche grazie all'Italia, all'energia, alla competenza dimostrata dal Governo, in particolare del ministro D'Alema, che hanno in qualche modo trascinato, per non dire obbligato, gli europei a muovere, in *primis* la Francia, che del Libano si voleva storica protettrice. Non è purtroppo infrequente che l'Italia sia presentata negativamente all'opinione pubblica Ebbene, il ruolo di guida ispiratrice che essa invece ha saputo giocare in questa occasione le è meritatamente valso un coro di elogi *in* *primis* proprio dalla Francia. L'Italia e altri Paesi europei hanno dimostrato particolare competenza già nella fase della negoziazione della risoluzione 1701, in particolare per quanto riguarda le regole di ingaggio, questione fondamentale perché una parte del discredito di cui è vittima l'ONU deriva proprio dal fatto che i caschi blu non dispongono spesso di istruzioni chiare e finiscono per ciò per essere più ostaggi o semplici e tragici spettatori che attori efficienti e convinti. Grazie anche principalmente all'Italia è stata costituita una missione certo di pace, ma adeguatamente organizzata, non disposta a farsi umiliare come accadde invece alle forze ONU nell'ex Jugoslavia, il che portò successivamente alla necessità di un intervento NATO al di fuori del quadro ONU per mettere fine alla follia nociva omicida di Slobodan Milosevic. Non è perciò abusivo sostenere che al necessario recupero di autorevolezza dell'ONU, solo antidoto all'anarchia internazionale e al rischio di guerre senza fine, si giungerà tramite missioni come quella che l'Italia si prepara a comandare. Nel dichiarare perciò il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento in oggetto e nell'augurare un pieno successo della missione, mi permetto solo un appunto. Serietà, abilità, lavoro silenzioso e attento hanno permesso di organizzare questa missione e di dare, come sottolineavo, un esempio al mondo. Non parrebbe saggio sciupare in parte il risultato esagerando o deformando l'aspetto mediatico del fatto. Devo inoltre sottolineare la necessità assoluta che la missione sia accompagnata da iniziative politiche e diplomatiche insieme con i *partner* europei, che devono rimanere il perno di tutta la missione. Abbiamo apprezzato la serietà, il realismo dei ministri competenti, Parisi e D'Alema, e soprattutto la convergenza di forze politiche della maggioranza e dell'opposizione, pur con i distinguo, le riserve, le preoccupazioni e le legittime motivazioni e posizioni di ognuno. Vogliamo esprimere ottimismo per la missione italiana in Libano, ma anche in questo caso ricordiamoci cosa vanno a portare i nostri soldati: non protagonismo, non avventura, ma un grande contributo alla pace in Libano e, più in generale, in Medio Oriente.

Il nostro sostegno non è certamente dato a cuor leggero, perché siamo coscienti di quanto tutta l'operazione sia complicata, complessa, non priva di rischi e anche di improvvise modifiche sul campo,

con prudenza e solo se unicamente rispondenti ad una serie di requisiti: il chiaro mandato ONU; un profilo certo di interposizione, di *peacekeeping* e, in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione (questo sì), la congruità

siamo lì con il consenso delle parti in causa, fatto estremamente importante e da sottolineare. Ma questa missione, lo voglio ribadire con forza, è in assoluta discontinuità con le missioni precedenti in Iraq e Afghanistan. Troviamo quindi, lo dico con estrema franchezza, assolutamente pretestuoso e strumentale, come si è visto nel dibattito di prima sugli ordini del giorno, il tentativo di rappresentare la missione in Libano in continuità con le scelte del precedente Governo.

subito dopo, così come è stato in Iraq, una guerra decisa al di fuori dell'ONU, in violazione del diritto e della legalità internazionali, o come è stato per la missione in Afghanistan, che seguì l'intervento unilaterale degli Stati Uniti, coperta solo *ex post* da una risoluzione del Consiglio di sicurezza. Quindi, vi è una bella differenza con l'impegno di oggi in Libano che nasce, invece, per interrompere una guerra, mettere fine alle sofferenze della popolazione, contribuire a ristabilire la statualità e la sovranità piena del Governo libanese e soprattutto, in prospettiva, costruire un percorso di pace in tutta la regione. Nazioni Unite è chiarissima a questo proposito nell'indicare come uno degli obiettivi del contingente ONU e della missione l'aiuto al Libano per ricostruire la propria statualità e sovranità sull'intero Paese come sia centrale anche l'aiuto alla popolazione civile. In questo quadro, è altrettanto chiaro che la missione UNIFIL 2, per quanto riguarda il disarmo di Hezbollah vice ministro Intini è stato chiarissimo), che è certamente una delle cause delle tensioni fra Israele e Libano, non ha né potrebbe avere il compito di intervenire direttamente, ma solo attraverso l'aiuto allo Stato libanese a ristabilire la propria sovranità all'interno dei confini. evidenzia le difficoltà che si incontreranno nell'applicare il vero punto, che è politico e diplomatico, nel dare una soluzione alla questione; questo punto non è certo costituito solo e unicamente dal dispiegamento dei contingenti militari, ma piuttosto dall'inizio di un nuovo processo politico e diplomatico che stabilisca nuove regole di convivenza fra i due Paesi e in tutta l'area. Il nostro Paese si è speso a livello internazionale e in Europa per tale missione, proprio per dare l'avvio ad un percorso di pacificazione e di pace. È qui il segno nuovo e di discontinuità con la politica estera del Governo precedente. È l'inizio di un nuovo corso, certamente non automatico, non scontato, non semplice della politica internazionale dell'Italia, che riprende il suo storico ruolo diplomatico con i Paesi mediterranei e i Governi arabi, che però può essere il segno di un nuovo corso delle relazioni internazionali. Soprattutto, non posso non sottolineare che, grazie all'iniziativa forte e determinata del nostro Paese (a cominciare dalla Conferenza di Roma), finalmente anche l'Europa, assumendosi le proprie responsabilità, è ritornata in campo per giocare - speriamo - un ruolo forte

Dopo cinque anni di svuotamento e mortificazione dell'ONU, di unilateralismo statunitense, di guerra infinita e preventiva, che ci ha consegnato un aumento a dismisura del terrorismo e dell'insicurezza dei nostri Paesi, tragedie umanitarie e guerre civili come in Iraq (altro che democrazia), forse si può riaprire una nuova stagione di multilateralismo che rimetta al centro delle relazioni internazionali il diritto e la via della diplomazia, della cooperazione e del dialogo. Il Libano è un banco di prova per capire se il nuovo corso è reale, se ha le gambe per camminare, se la nuova stagione di multilateralismo si può davvero aprire. Per tale motivo, ci preme sottolineare che la missione UNIFIL 2 non è la conclusione di un percorso, perché la presenza militare è solo di aiuto (anzi riteniamo sempre più che bisognerà porre l'accento anche sulla parte della cooperazione civile)

causa dei conflitti continui di tutta l'area. Qui devono tornare in campo i processi politici; qui si può misurare il nuovo corso; qui gli elementi positivi del cambio di passo della politica internazionale debbono registrare un'efficace ricaduta affinché davvero si lavori perché dalla crisi libanese si possa riprendere un percorso per arrivare ad una conferenza di pace in Medio Oriente

Per questi stessi motivi, nell'accingerci ad esprimere un voto favorevole alla missione, vorremmo ancor di più che il cambiamento della politica internazionale del nostro Paese,

è necessario riflettere seriamente su tale missione. Siamo ancora in attesa di capire che fine ha fatto il monitoraggio, ma, soprattutto dopo l'ulteriore drammatizzazione della situazione in Afghanistan, credo sia nostro dovere indicare chiaramente la via del disimpegno delle nostre truppe da quel contesto, tanto più oggi che il nostro Paese ha necessità di concentrarsi in Libano. Il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani voterà dunque a favore della partecipazione alla missione in Libano, nella speranza che essa ponga le basi di un vero processo di pace. Ciò potrà accadere solo e unicamente se il nostro Paese, insieme con l'Europa e l'ONU, sapranno dispiegare, oltre che un contingente militare, una forte azione diplomatica e costruire in quelle terre martoriate ponti di pace, ritessendo il filo del dialogo che anni di odio e e terrore sembrano aver spezzato. Oggi pensiamo che anche con l'ingresso dell'Italia nel Consiglio di sicurezza la strada può forse apparire meno faticosa e in salita.

che autorizza la missione in Libano. Questa scelta è stata fatta dal nostro Gruppo sin dal primo momento, in omaggio e in coerenza alla propria tradizione politica e al convincimento che la politica estera, quando possibile, debba rappresentare un bene comune del Paese e del Parlamento e che perciò sulla politica estera, quando possibile, sia preferibile evitare divisioni strumentali. Tuttavia, proprio il dibattito svolto nell'Aula del Senato, ancor più è diversamente dal dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, ha dimostrato ed evidenziato talune ombre dalle quali il nostro atteggiamento non rimarrà condizionato, ma che è opportuno mettere invece in luce. Le motivazioni con le quali alcuni Gruppi parlamentari convergono sul voto favorevole alla conversione del decreto-legge del decreto-legge sono contrastanti e antitetiche alle motivazioni esposte con estrema chiarezza dalla relazione introduttiva, nei confronti della quale esprimo apprezzamento, svolta dal senatore Polito e peraltro ribadita dall'intervento del presidente della Commissione difesa, senatore De Gregorio. L'Italia va in Libano per una missione di pace, ma lo fa nel quadro di una risoluzione ONU, la 1701, ONU, la 1701, in cui si fissano con molta chiarezza gli obiettivi: ripristinare la pienezza dell'autorità e della sovranità dello Stato libanese; assicurare certezza ai confini di Israele. Orbene, non bisogna dimenticare che la crisi di luglio non è stata determinata da un'improvvisa insorgenza bellicista di Israele, ma l'azione di Israele è stata la conseguenza di provocazioni, che hanno avuto un episodio specifico nel rapimento di due soldati israeliani, ma che hanno un retroterra molto consistente. Il punto che sarà al centro di tutta l'attività e anche della possibilità di successo e di riuscita della missione di pace è costituito dall'attività degli Hezbollah. È bene, onorevoli senatori, non sfugga all'attenzione di alcuno che il rischio fondamentale per la missione in Libano è rappresentato appunto dalla possibilità che gli Hezbollah

punto di sfida, che evidentemente andrà affrontato e risolto politicamente. Orbene, credo di non dover dire cose che sfuggano all'attenzione di alcuno di noi e ritengo che su questa materia il confronto debba avvenire sempre con molta franchezza. Gli Hezbollah sono un gruppo terroristico che non è autonomo rispetto al quadro del terrorismo quale esso è, o determinato, o ispirato, o sollecitato, o guidato da almeno due Paesi, Siria ed Iran. ed Iran. Il punto di successo diventa allora un punto politico. È o sarà possibile indurre la Siria e l'Iran ad accettare definitivamente

Israele? Se non si ottiene questo risultato per le vie politiche, allora la missione di pace, che sino a questo momento ha sortito un risultato che tutti dobbiamo apprezzare, cioè una tregua, otterrà che questa tregua sia soltanto provvisoria e transitoria. Credo che ognuno di noi debba sforzarsi di augurare a questa missione il successo. Ma mi permetto di osservare che, quando si sottolinea con particolare enfasi l'aspetto europeista - il senatore Zanone richiama sempre questa caratteristica, che la missione stessa avrebbe assicurato attraverso l'iniziativa italiana e quando penso (e mi lascio sovrastare da questa preoccupazione) che a febbraio il comando della missione passerà dalla Francia all'Italia, io sono tentato di avanzare un cattivo pensiero, cioè che i francesi vogliano lasciare il comando all'Italia nel tempo in cui la situazione in Libano potrebbe essere diventata molto difficile. Infatti, o entro febbraio, autonomamente e volontariamente, gli Hezbollah si politicizzano e abbandonano le armi, oppure c'è il rischio elevatissimo che gli Hezbollah, con l'arsenale che probabilmente in queste settimane hanno ricomposto, senza che sino a questo momento ci sia stata dalla missione di pace UNIFIL alcuna interposizione significativa, effettiva ed efficace, minaccino ancora una volta Israele. È a quel punto che le truppe impegnate in Libano potrebbero correre un grandissimo rischio. È stato invocato e richiesto molte volte che si precisi articolatamente quello che io chiamo il regolamento di servizio, cioè la regola di ingaggio. Orbene, la regola di ingaggio dimostrerà tutta la sua debolezza in quella fase ed in quel passaggio. È questa preoccupazione che deve indurre il Governo italiano a proseguire nell'iniziativa che ha intrapreso, non già per rivendicarne i meriti. Ascolto sempre con molta attenzione il senatore Tonini; però oggi ho avuto un attimo di esitazione quando egli ha usato la parola «interventismo» e l'ha corretta nel suo significato, che le pagine della storia ci trasmettono in modo non certamente positivo, con un bell'aggettivo, parlando di «interventismo pacifista». Sarei molto prudente ad intervenire anche con intendimenti di pace, anzi ritengo che le due parole facciano a pugni tra di loro. Però, è possibile che l'Italia assuma anche una responsabilità maggiore di quella che avrebbe dovuto e di quella che avrebbe potuto. Il Governo non riceve la nostra critica e men che mai la nostra sanzione, anzi ha ricevuto dall'UDC sostegno in questa iniziativa, perché riteniamo che sia necessario l'Italia abbia una pienezza di responsabilità nelle politiche che tendono ad assicurare la pace nel quadrante mediorientale. Ma ciò non può minimamente giustificare alcuna enfasi come quella che è stata ripetuta molte volte anche in quest'Aula questa sera. Allora, il consenso che diamo alla conversione del decreto‑legge, onorevoli senatori, è politicamente politicamente motivato, ma è un consenso - uso delle parole precise - che diamo con timore e con tremore, per utilizzare le parole di Romano Guardini.

pur tuttavia che anche per noi non è facile ogni volta vedere l'utilizzo dello strumento militare. Però, in questo caso ci sembra che sia nel quadro della legalità internazionale, soprattutto per aprire uno spazio di trattativa, uno spazio alla diplomazia internazionale in cui il nostro Paese si sta già molto adoperando e bene. Ribadisco il nostro voto favorevole, con l'auspicio che

Presidente, nel corso di questo dibattito - siamo anche un po' amareggiati - non abbiamo visto né sentito, non si è avuto sostanzialmente neanche il pudore di sostenere delle posizioni corrette. Nessuno, per esempio, ha avuto la correttezza di ammettere una minima verità; non si è né saputo, né voluto ammettere infatti, che anche le altre missioni rispettavano l'articolo 11 della Costituzione; tutte le missioni hanno avuto un supporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Altrimenti - e questo lo diciamo alla maggioranza - anche il loro rifinanziamento, appena votato alcuni mesi fa, avrebbe colliso con l'articolo 11 della Costituzione. Un altro aspetto: abbiamo un grosso timore che si vada verso il riarmo dei terroristi di Hezbollah. Quali sono le motivazioni?

Noi sappiamo, per esempio, che il Governo centrale libanese non ha il controllo del territorio; sappiamo di più, che tollera la presenza di formazioni militari irregolari su quella parte di territorio. Queste armi in quali mani finirebbero? Terzo problema che ci rammarica è che probabilmente è finita la campagna contro il terrorismo internazionale alla quale anche l'Italia ha aderito all'indomani dell'11 settembre 2001. ci sembra un po' affievolita la nostra posizione nei confronti dei terroristi, sembra più che l'Italia o il Governo italiano volesse intervenire quasi in modo punitivo nei confronti di Israele, piuttosto che disarmare i terroristi. L'ultima questione che lascia molto perplessi è la visita di Prodi in Libano all'inizio del mese di ottobre: non solo è stato ricevuto con il benvenuto degli alti dirigenti di Hezbollah, ma ha avuto anche i ringraziamenti da questi per la tolleranza che i nostri militari e tutto il contingente UNIFIL avrebbero nei confronti delle milizie irregolari. Tolleranza: vuol dire che le armi non si vogliono assolutamente vedere. A questo punto, signor Presidente, non capiamo quale sia l'obiettivo del Governo italiano in questa missione:

libanese. La Lega non può e non è d'accordo nel mandare i propri ragazzi a combattere con regole oscure, del resto col codice militare di pace, mentre gli altri contendenti sono in guerra;

Signor Presidente, riprendo le parole del collega Mannino: ci apprestiamo a votare a favore di questo decreto-legge con molto timore e con molti tremori, che sono anche emersi in molti interventi della maggioranza, a cui va dato atto di una elevata onestà intellettuale che abbiamo registrato oggi nel dibattito. Ma il timore e il tremore si accompagna anche a un'enfasi che questo Governo sta mettendo alla politica estera e ai fatti di politica estera che altrettanto ci preoccupano. Vorrei citare un esempio che non ha attinenza a quello del Libano, ma che è di attualità. Noi non possiamo che essere soddisfatti del risultato conseguito ieri e dell'ingresso dell'Italia nel Consiglio di sicurezza; ci pare strano, però, che questo avvenga in un clima per cui il Presidente del Consiglio dice che è un fatto storico: forse gli dovreste spiegare dalla Farnesina che non è la prima volta che entriamo nel Consiglio di sicurezza, così come forse dovreste spiegare che nel 2001 chiedemmo di entrare nel Consiglio di sicurezza e fummo battuti perché le regole dell'avvicendamento allora non ci vedevano in grado di entrare in questo consesso. Voglio ricordare che questa candidatura è stata posta nel 2003 e allora forse, senza usare parole mie, ma citando le parole di un famoso ambasciatore che ben conosce l'ONU, Francesco Paolo Fulci, credo valga quanto oggi si dichiara sul «Corriere della Sera»: «il merito del nostro successo va sia al Governo Berlusconi, il quale stabilì un rapporto speciale con l'Amministrazione Bush, sia al Governo attuale, che ha ribadito l'impegno in Afghanistan e ne ha assunto uno nuovo in Libano, sia al lavoro costruttivo della diplomazia al Palazzo di vetro e sul campo nel corso dei decenni». E forse qui mi coglie l'occasione di rivolgere un sincero ringraziamento alla diplomazia italiana e al suo capo, l'ambasciatore Spatafora, che ha guidato brillantemente quest'operazione. Ma anche quando si cita questo successo, misurato in 186 voti, che certamente è un risultato apprezzabile, voglio ricordare che il Sudafrica ha ottenuto la stessa votazione e che l'unico vero obiettivo che abbiamo raggiunto - e di questo siamo soddisfatti - è quello di avere battuto il Belgio che ne ha presi 180 e quindi possiamo dire di avere vinto sei a su un fatto così rilevante, sul quale certamente tutte le forze politiche del Parlamento non possono che esprimere soddisfazione, vi è un'enfasi da parte del Governo che francamente ci preoccupa, perché qualche volta ci sembra dagli interventi anche del Governo che l'ONU sia stato inventato dopo l'11 aprile e che il multilateralismo sia una proprietà di questo Governo e non una storia continua della politica estera italiana; così come ci stupisce che lei stesso, vice ministro Intini, abbia usato all'inizio del suo intervento un preciso riferimento a tre pilastri della politica estera nazionale: l'Unione Europea, la NATO e l'ONU, e non è la prima dichiarazione ufficiale del Governo; quando vi si chiede di articolare in un documento parlamentare la stessa valutazione che fate in quest'Aula, riceviamo una risposta assolutamente negativa. Questo è un altro aspetto: è come se questa enfasi del enfasi del multilateralismo fosse una proprietà indivisa da parte del Governo di centro-sinistra e non una storia continua e un riferimento preciso della politica estera italiana.

Qualche conoscenza l'abbiamo in materia. Sull'argomento esiste una lettera dell'ex ministro degli esteri Shara, attuale vice presidente, al segretario del generale dell'ONU nella quale si dice che loro avrebbero trattato regolare con il Libano l'eventuale appartenenza territoriale di queste fattorie. Sostenere oggi che si chiede che Shebaa venga liberata dalle truppe israeliane passa per un altro assioma, quello per il quale Hezbollah sostiene di essere una grande forza nazionale libanese e che resterà in armi fin quando non verranno restituite le fattorie di Shebaa. Pertanto, può anche trattarsi di carattere geografico, ma mi preoccupa un'enfasi che forse nasconde un *lapsus* di carattere politico, e quindi di un apprendimento di Hezbollah che ormai è entrato nella vicenda. Francamente devo riconoscere di essere rimasto perplesso da questo conteggio matematico sul costo dell'operazione e sulla diminuzione del prezzo del petrolio. Credo che sia molto difficile misurare la pace in termini di prezzo del petrolio.

le giuro non dall'opposizione, ma credo dal suo Presidente del Consiglio, il quale forse non ritiene di dare alla politica estera quell'autonomia che, devo dire giustamente, la Farnesina aveva chiesto almeno per non combinare sempre un discorso di carattere economico-finanziario rispetto a un argomento politico evidentemente prevalente. Il fatto che in questa strana mediazione forse significa che avrete mal di pancia una volta l'anno invece di due quando tratteremo dell'Afghanistan, ma non abbiamo risolto un problema di ben altra natura e livello, essenzialmente di carattere politico. Ma tremori e timori vengono non tanto per le regole d'ingaggio. Anche qui, liberiamoci da qualche ipocrisia: non credo succederà mai che l'esercito libanese chieda alle truppe italiane dell'UNIFIL di andare a disarmare Hezbollah. Questo è un pericolo che non esiste e ne siete assolutamente coscienti. *(Applausi del I tremori e i timori vengono pertanto da un'altra valutazione, che l'onestà intellettuale del collega Tonini oggi ha posto all'attenzione dell'Aula. Questo è un intervento militare ad altissimo livello politico, proprio seguendo la vostra impostazione. Questo è un intervento che va a porre una forza di interposizione. Onestamente abbiamo ottenuto un successo: abbiamo fatto cessare la guerra. Ma questo tampone, la forza di interposizione, ha un valore e un significato se la sua durata è breve, se riesce a dare in tempi necessari un'azione politica che possa modificare le ragioni per le quali UNIFIL è intervenuta. Altrimenti la missione UNIFIL 2 diventerà la copia di UNIFIL 1, che ricordo essere in quelle zone dal 1978 e che non ha assolutamente ottenuto nessun risultato: prova ne sia che Hezbollah dichiara ancora oggi di aver 20.000 missili che - come lei ben sa, signor Vice Ministro anche se è accertato dai bombardamenti israeliani che tutti i depositi di Hezbollah sono vicini alle sedi della stessa UNIFIL 1. Infatti, come spesso capita e a vecchi latitanti siciliani e sardi insegnavano, il posto migliore per rifugiarsi è la caserma dei carabinieri. Con questo principio, lo stesso dei latitanti sardi e siciliani, Hezbollah ha operato e la missione UNIFIL 1 non ha visto assolutamente niente. il problema su cui chiedevamo una risposta al Governo e su cui ci aspettavamo, dopo l'intervento del ministro D'Alema in Commissione, che qualche risposta ci arrivasse (ha ragione il collega Selva a dire che attende una risposta dal Governo per sentirsi liberato da un voto che lo preoccupa) è quello di rivelare, visto che ci siamo impegnati con 3.000 uomini a un costo di 100 milioni di euro al mese e abbiamo impegnato l'immagine del nostro Paese in una situazione rischiosa, l'obiettivo politico che il Governo si pone. Qual è il valore aggiunto d'iniziativa politica che il Governo italiano - insieme all'Europa, certamente, perché essendo voi multilaterali giocate in squadra - deve ottenere? Quali sono le novità? La Siria e l'Iran? Forse. Nessuno si scandalizza, soprattutto di un rapporto diverso con la Siria. Ma quale e in che modo? Cos'ha oggi l'Italia da giocare su questa carta internazionale? Visto che siete europeisti, vi ricordo che l'inizio della frattura con la Siria avvenne per la mancata firma del trattato di associazione della Siria all'Unione Europea. Non fu la Siria a rifiutarsi di firmare, ma l'Unione Europea che, condizionata dalla sua politica, non arrivò a sottoscrivere quel trattato che avrebbe forse consentito un'evoluzione del regime siriano verso forme molto diverse da quelle che conosciamo

in dissenso è un dato meramente tecnico per poter parlare con rispetto della posizione che il mio partito ha assunto, ma con eguale rispetto per le mie convinzioni e, soprattutto, per via del fatto - mi rivolgo al vice ministro Intini - che nessuna delle domande da me poste questa mattina ha trovato nella sua replica una risposta. concerne una missione che il Ministro della difesa ha definito lunga, difficile e rischiosa, noi non sappiamo, ad un mese e mezzo dall'inizio, come si stia svolgendo.

cui la scoperta delle armi possedute dagli Hezbollah sia affidata ai libanesi (come sappiamo), questi non

Si tratta, come peraltro il Governo ha detto più volte, di una missione impegnativa, costosa e rischiosa, per questo avremmo preferito, come del resto aveva detto il Ministro degli esteri dinanzi alle Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato, che il Governo tenesse costantemente informato il Parlamento. Lo stesso Ministro, di fronte alle Commissioni, ha dichiarato che in quel momento non c'era un mandato in bianco del Parlamento al Governo, ma si stavano svolgendo degli atti preparatori e poi ci sarebbero state delle delibere successive. Ciò non è avvenuto (il ministro D'Alema, a dir la verità, non è nuovo a questo comportamento e basta, a tal proposito, ricordare la missione in Kosovo). Un maggiore coinvolgimento del Parlamento da parte del Governo, sarebbe stato più consono, anche perché questa missione, come dicevo, è piena di complessità e difficoltà. Anche le recenti affermazioni di Nasrallah, devono farci preoccupare: «Hezbollah» - egli afferma - «dispone di notevoli quantità di missili e razzi (...) Non si lascerà disarmare perché si farebbe il gioco dei sionisti». Sono affermazioni molto gravi, perché con questi atteggiamenti si continua a non ottemperare alle risoluzioni ONU, perché sono armi che possono essere utilizzate contro le popolazioni civili israeliane, perché è la premessa per un nuovo possibile conflitto. Tutti sappiamo che l'esercito libanese non ha la possibilità di operare per azzerare gli arsenali Hezbollah. Da qui, la preoccupazione. Anche per questi motivi, sottolineiamo le difficoltà della missione militare: difficoltà per lo svolgimento dell'UNIFIL 2, che non deve ripetere gli esiti di UNIFIL 1, che indubbiamente ha consentito a Siria e Iran di armare Hezbollah, componente palesemente terroristica; difficoltà per i nostri militari e per i rischi evocati da sempre, anche per le perplessità e le incertezze delle modalità operative. In questo senso, la missione corre il rischio di dare tempo a una ricostruzione degli arsenali Hezbollah, che potrebbero continuare a costituire un grande pericolo per Israele. Da qui, la necessità di sviluppare una più forte azione di politica internazionale per bloccare le azioni e le attività di Siria e Iran. Credo che questo sia un impegno importante, da parte nostra,

ma disponibilità di tempo per un processo di pace che dia sicurezza a Israele e stabilità al Libano. Infatti, la situazione in Libano costituisce, come dice la risoluzione, una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Da qui la nostra responsabilità, perché dobbiamo esprimere un voto favorevole un voto favorevole e dare tempo all'azione politica internazionale per la quale chiediamo al Governo di assumere una posizione urgente e forte, ma equilibrata. Non riteniamo - signor Presidente, ho quasi finito che per questioni di equilibri interni della maggioranza ci sia la continuazione di un atteggiamento e di un posizionamento che appare più contrario a Israele e più favorevole a una posizione Hezbollah. Certe passeggiate inevitabilmente suffragano questo segnale. Dobbiamo e vogliamo dare solidarietà ai Paesi arabi moderati e ad Israele, la cui sicurezza sarebbe fortemente messa in forse da un riarmo Hezbollah. Hezbollah. Concluderò dicendo che vogliamo dare un segno di continuità della nostra politica estera, che sulla base dei grandi pilastri delle Nazioni Unite, dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica ha sempre visto il nostro Paese in una posizione di grande impegno internazionale in operazioni di pace e di sviluppo e di concordia tra i popoli. Posizione di continuità ed impegno che ci viene riconosciuta internazionalmente. A distanza di un decennio, ritorniamo nel Consiglio di sicurezza per il prossimo biennio: non è un episodio contingente, facilitato, come dice il vice ministro Intini, dalle ultime decisioni del Governo italiano. Ci sono motivi seri e forti, che sono l'impegno internazionale dell'Italia. Dicevo - e concludo - che questa nostra posizione di grande responsabilità non deve essere considerata come un mandato in bianco, indefinito nel tempo, da parte nostra nei confronti del Governo. Desideriamo che il Governo, costantemente, tenga informato il Parlamento sull'andamento della missione, sulla impostazione operativa, sulle attività e gli atteggiamenti politici. Desideriamo che ci sia una costante verifica. Dobbiamo essere sicuri e certi che, pur nell'ambito dei rischi insiti in ogni missione militare, i nostri soldati non debbano venirsi a trovare in condizioni di difficoltà o di essere ostaggio di nessuno. Dobbiamo evitare che nessuno guadagni tempo per destabilizzare ulteriormente quell'area così delicata. Concludo, ribadendo che il voto è favorevole per ragioni di solidarietà internazionale nei confronti dei Paesi arabi moderati e di Israele, che possono trarre giovamento da questa missione, per la vicinanza e un segnale di unità di tutta la Nazione ai nostri militari che sono internazionalmente apprezzati per il loro impegno, la loro capacità e umanità nelle missioni e a cui non toglieremo mai la nostra copertura;

assolutamente convinto e direi felice di votare no, un no assoluto, totale a questa missione, dopo aver ascoltato tutti gli interventi - a cominciare da quello del Governo, del vice ministro Intini - che dimostrano come ci sia una rottura totale nella linea della politica estera italiana. Questo lo dico ai miei colleghi, della mia parte politica, che hanno usato con me, nelle nostre discussioni, tale argomento: non si può assolutamente dissentire, quando è in gioco la politica estera del Paese. Ebbene, questo presuppone che esista una forma di continuità. di continuità. L'abbiamo vista! Il seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed il prestigio, di cui si è avvalso questo Governo per portare avanti l'azione sul Libano certamente non nascono da pochi giorni di Governo, ma dal prestigio di un Governo precedente, il quale ha agito sul piano internazionale in maniera forte e determinata. Su questo si è basato il successo internazionale diplomatico. *(Applausi dal Gruppo FI).* Questo successo è stato poi usato

parliamo magari del Governo di Haifa; uno non dice il Governo di Washington o il Governo di Parigi!). Inoltre vi do una notizia: le agenzie di stampa del Medio Oriente hanno lanciato una

missili aria-terra che possono colpire gli aerei israeliani. Ricordo che precedentemente la fregata israeliana è stata colpita da un missile di fabbricazione cinese, importato dall'Iran, impostato su un *radar* dell'esercito libanese, che contiene Hezbollah al proprio interno. Questa missione va a sostenere Hezbollah. Questa missione va a colpire gli interessi della pace in Medio Oriente e a non risolvere alcun problema. Ed è molto grave che la parte politica della Casa delle Libertà non l'abbia capito e si accodi nella sua maggioranza ad una decisione sbagliata e sciagurata.

sfugge che la missione in Libano è al contempo difficile e rischiosa, ma anche occasione di opportunità per la soluzione dei problemi più generali dell'area del Medio Oriente. Ed è stato, utile quindi, che il dibattito si sia svolto in un clima, tutto sommato, sereno e costruttivo come già avvenuto alla Camera. Ma non posso fare a meno di notare, rispondendo ad alcune polemiche di qualche collega dell'opposizione, che nella fase di votazione degli ordini del giorno e, soprattutto, degli emendamenti presentati da una parte dell'opposizione, la stessa si è divisa in più parti. L'Italia è stata tra i Paesi che hanno promosso la missione ed è il Paese che ne assumerà la direzione tra qualche mese. Siamo, quindi, responsabilmente impegnati in maniera rilevante e non soltanto per la consistenza dell'apparato militare. E quindi spiace che nelle parole del senatore Mantica, collega che stimo e non da oggi, si banalizzi in questo momento, dopo averla definita prima troppo ambiziosa e ai limiti dell'avventatezza, l'iniziativa diplomatica del Governo, sviluppatasi sin dalla Conferenza di Roma e con il lavoro diplomatico successivo, che ha avuto un rilevante peso nella risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza. Essa ha contribuito, in modo decisivo, a fermare il sanguinoso conflitto israelo-libanese e ad impegnare la comunità internazionale, ed in particolare l'Unione Europea, nell'avvio di un processo teso a ridurre la conflittualità di un'area cruciale della regione mediorientale e di un'area che si trova nel cortile di casa nostra. È sicuro che il Medio Oriente necessiti di una soluzione globale, perché non esistono soluzioni parziali ai problemi complessi presenti in quell'area: da qualche parte, però, bisogna pur cominciare. Certo, si deve procedere gradualmente, si deve creare un contesto internazionale e territoriale che consenta di affrontare e di risolvere con risposte durature e definitive un gravame di questioni che si trascinano da oltre 60 anni. Taluno ha sottolineato di non volere una missione che si svolga in un contesto ambiguo di politica estera: è giusto. Infatti, in questo caso, discutiamo di una missione stabilita in sede Nazioni Unite, sostenuta dal nostro principale alleato, gli Stati Uniti d'America, che da anni - come avviene per altro anche nell'ambito dell'Alleanza atlantica - chiede chiede un maggiore impegno del pilastro europeo nelle missioni internazionali di pace. La missione è sostenuta anche dall' Unione Europea ed a ed a seguito della deliberazione del 18 agosto scorso - va detto in quest'Aula - ha avuto ampio sostegno da parte dell'intero arco politico, di maggioranza e di opposizione, salvo l'astensione della Lega su un parte di quella risoluzione. Dunque, abbiamo un contesto di politica estera chiaro, più condiviso sul piano sia internazionale che nazionale di quanto non sia stato per altre missioni. L'Europa, divisa sulla guerra in Iraq, in occasione della crisi libanese ha conosciuto una sorta di riscatto, di assunzione di responsabilità e di ruolo. Determinante è stata l'iniziativa dell'Italia, dalla convocazione del Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione Europea alla presenza di Kofi Annan, all'assunzione della principale responsabilità nella costituzione della UNIFIL rafforzata. L'elezione dell'Italia al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con voto pressoché unanime dell'Assemblea delle Nazioni Unite, mette il sigillo al riconosciuto valore aggiunto che la nostra politica estera apporta alla gestione delle più delicate problematiche della comunità internazionale. Ecco perché, dopo un fatto di così rilevante significato per tutta l'Italia, non solo per la maggioranza, francamente non appassiona l'ennesima discussione sulla vicenda irachena. Credo che dobbiamo piuttosto mettere l'accento su un dato: alla base della nostra politica estera concorrono i tre pilastri fondamentali cui spesso anche in questo dibattito si è fatto riferimento: le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'Alleanza Atlantica. Bene: alla missione in Libano concorrono tutti e tre questi cardini. Si tratta, infatti, di una missione stabilita in sede ONU, appoggiata dagli Stati Uniti e sostenuta dall'Unione Europea. Questa nuova soggettività dell'Europa ha certamente contribuito ad una diversa considerazione dell'amministrazione degli Stati Uniti nei confronti del multilateralismo, anche grazie alla linea di azione politico-diplomatica che l'Italia ha efficacemente perseguito riavviando il dialogo con tutti i soggetti politici e istituzionali rilevanti nel Medio Oriente. In sostanza, la capacità del nostro Paese di porsi come interlocutore credibile e affidabile di tutte le parti in causa è un patrimonio utile al riaprirsi di un processo di pace in Medio Oriente e dunque al dialogo tra tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in un'epoca nella quale il fondamentalismo di matrice terroristica persegue viceversa il conflitto di civiltà. Un coraggioso uomo di Governo israeliano, di fronte alle contestazioni della politica del dialogo sviluppata da Israele e alla scommessa della pace, rispose che «la pace si fa con i nemici, perché con gli amici è un dato di fatto». Questa è la migliore risposta alle perplessità espresse da alcuni rispetto ad un necessario dialogo anche con l'Iran e la Siria. del resto, con l'Iran sul nucleare già ha luogo da tempo. Si deve trattare naturalmente di un confronto basato su elementi di chiarezza, senza dare luogo a cedimenti o a suggestioni distorte. La pace deve essere un fatto vero e basarsi su una composizione vera degli interessi, ad iniziare dal diritto del popolo d'Israele e della Palestina a vivere in pace entro confini internazionalmente riconosciuti. Trattare significa anche sottrarre l'interesse dei palestinesi ad avere il loro Stato ostaggio di tutti gli altri interessi dell'area. Quindi, facciamo qualcosa oggi, ma in una prospettiva di più lungo termine, gettando un seme che può produrre risultati ben più solidi ed ampi dei compiti della missione UNIFIL. Raggiungere un rafforzamento reale dello Stato libanese, della sua sovranità, della sua autonomia; porre fine al persistere di milizie armate, al di fuori della propria autorità e del proprio controllo; conseguire, attraverso le vie della politica, del dialogo e della diplomazia, una ridefinizione del ruolo della Siria e dell'Iran nel contesto regionale: sono obiettivi qualificanti, possibili e utili, perché quello che è avvenuto questa estate è un accenno del grande fuoco che potrebbe divorare l'intera area. Il successo della missione contribuirà in modo rilevante a riaffermare e difendere il diritto dello Stato d'Israele a vivere in sicurezza e in pace entro i propri confini, collegando così questa missione con il più ampio problema degli equilibri della convivenza pacifica nell'insieme della regione. Per questa serie di ragioni, che ho fin qui succintamente esposto, sosteniamo con convinzione la partecipazione italiana alla missione UNIFIL 2, sia per ricostruire tutti gli elementi che permetteranno al Libano di avere un ruolo all'interno di un sistema multiconfessionale e multietnico, sia per aprire la porta al dialogo e alla pace in tutto il Medio Oriente.